la legge finanziaria sulla quale è stato posto il voto di fiducia, mostra innumerevoli contraddizioni: in ordine alla politica fiscale e alla situazione delle entrate che si è manifestata nell'anno in corso, alla destinazione delle risorse e all'innumerevole mole di norme contenute, alla corrispondenza rispetto al Documento di programmazione economica e finanziaria e al programma elettorale con cui l'Unione si era presentata agli elettori. Trattare di tutti questi aspetti non mi è possibile, per i tempi di cui dispongo, ma la consistente componente fiscale, e più in generale delle entrate, ritengo meriti un approfondimento. Infatti, un bilancio pubblico che dispone di impreviste e positive maggiori entrate che variano da un minimo accertato di oltre 33 miliardi di euro ad un massimo, da verificare entro la fine dell'esercizio, di circa 38 miliardi, non può in maniera imperterrita conservare nella programmazione per il 2007 una manovra di 34,3 miliardi, composti per due terzi dalle maggiori entrate dovute all'aggravio della pressione fiscale o, perlomeno, non lo può fare senza causare un rallentamento dell'economia che si manifesterà nel 2008, determinando un'inversione di tendenza rispetto alla pur flebile ripresa dell'anno in corso. Non può esistere altra motivazione seria, se non quella ideologica, a giustificare un simile atteggiamento che si può riassumere nei seguenti princìpi elementari: in un contesto di elevata pressione fiscale, di elevato debito pubblico, finanziario e burocratico, di ciclo recessivo, come detto, solo recentissimamente e minimamente convertito in un ciclo di crescita, di sottocapitalizzazione industriale, di *gap* tecnologico e d'investimento, il bilancio pubblico, a fronte di ottime e maggiori entrate fiscali, incrementa ulteriormente la pressione fiscale dello Stato e, indirettamente, degli enti locali, pur senza individuare concrete strategie e stanziamenti per favorire crescita, sviluppo e consumi. Oltre a questo, pur avendone correttamente individuato la pericolosa consistenza al tempo dell'approvazione del DPEF, non interviene a frenare la spesa pubblica corrente, vera spina nel fianco del bilancio pubblico, anzi, demagogicamente e fortunatamente senza concreta attuazione, auspica il suo incremento con i proclami di trasformazione di centinaia di migliaia di contratti del pubblico impiego da tempo determinato a tempo indeterminato. Premettendo che la politica delle entrate attuata in questo primo scorcio di legislatura si trova nel decreto Bersani-Visco, nel decreto fiscale collegato e nella presente legge finanziaria, uno degli argomenti addotti a giustificazione di questa suicida politica fiscale consiste nel recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. A parte che non sono due aspetti, evasione ed elusione, comparabili, credo sia interessante fare nel merito alcune considerazione sui recenti dati forniti dall'ISTAT sull'economia sommersa, per comprendere come, al contrario, il recupero dell'evasione così programmato sia solo una pia illusione. La relazione tratta correttamente del termine sommerso, attribuendo valore distinto alle varie componenti, precisando che nell'esame vengono identificate «le diverse «le diverse componenti della stima complessiva del valore aggiunto, riconducibili al fenomeno della frode fiscale e contributiva». Quei dati indicano che il valore aggiunto del sommerso

e mostra, nei dati storici, un modesto incremento tra il 2000 e il 2001 e un'interessante contrazione (tra 1 e 1,5 punti percentuali) dal 2001 al 2004. Ciò dimostra che l'evasione non è affatto aumentata nel quinquennio precedente, anzi è diminuita; ciò dimostra altrettanto che gli strumenti impiegati nel quinquennio precedente (anche i vituperati condoni, anche il rientro dei capitali a tassi vantaggiosi) non hanno creato aspettative di impunità. Anzi, la riduzione delle aliquote fiscali ha reso più appetibile il rispetto delle norme. Mettiamo una pietosa croce sulla pseudoredistribuzione equitativa dell'aggiornamento della progressività IRPEF attuata con questa finanziaria, da più parti dimostrata infruttuosa o negativa anche per i redditi modesti. Ma la relazione ISTAT è interessante anche per altri aspetti, ad esempio quelli riguardanti il sommerso stimato per le diverse aree di attività economica (con agricoltura e servizi che sopravanzano notevolmente l'industria) o quelli riguardanti le unità di lavoro, regolari o non regolari, per posizione nella professione (con i dipendenti che sopravanzano di gran lunga, tre volte e mezza, gli indipendenti). Questo ultimo dato non può che risultare ovvio - proporzioni contrarie non sarebbero ipotizzabili - però potremmo permetterci qualche riflessione su alcune gratuite criminalizzazioni fatte dal presidente del Consiglio Mi riferisco, in modo particolare, alle accuse di evasione rivolte all'artigianato e alla piccola impresa e alla tacita assoluzione di un variegato esercito, anche di dipendenti pubblici, che svolgono un secondo lavoro in nero. Se poi integriamo questi dati statistici con gli studi attuati sulla distribuzione territoriale dell'evasione, otteniamo un altro spaccato nei confronti del quale l'azione di repressione del Governo sarà assolutamente inefficace. Sul lavoro nero uno studio della CGIA di Mestre, rielaborando dati ISTAT, ha definito una tabella, con valori *pro capite*, che indica tra le Regioni più virtuose, nell'ordine, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana e, tra le più soggette al fenomeno dell'evasione, sempre a valori *pro capite* e nell'ordine, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Campania e Puglia. La domanda che mi pongo è allora la seguente: cosa è stabilito in finanziaria affinché il controllo del fenomeno trovi corrispondenza con l'individuazione di aree e settori a rischio? Nulla. Gli interventi e le norme sono indiscriminati; non esiste strategia legislativa ed operativa che conduca ad indirizzi specifici. Con il riferimento agli studi ISTAT ho voluto dimostrare che, alla vacuità propagandistica dell'azione fiscale della maggioranza e del Governo, corrisponde la concretezza penalizzante nei confronti di chi, invece, in gran parte adempie regolarmente ai propri doveri fiscali. Il motivo è molto semplice: se non si tiene conto né delle differenze settoriali né degli andamenti temporali né degli strumenti adottati in tali periodi né delle distribuzioni territoriali, quale risultato potrà essere ottenuto nella lotta all'evasione fiscale? Se invece, dietro al paravento della lotta all'evasione, si opera solo con strumenti che aggravano la burocrazia, con adempimenti minuziosi ed astrusi (tra i quali svetta, per ingegno, quello del pagamento con strumenti bancari dei professionisti), con la camicia di forza degli studi di settore, con l'inasprimento della curva delle aliquote, dell'incremento delle aliquote sulle rendite finanziarie, o con tutti i consistenti ritocchi utili a reperire nuove entrate (sulle autovetture, ad esempio, di uso aziendale), non si produrranno che crisi settoriali, contrazioni nei consumi, probabilmente maggiore evasione. Un esempio tra i molti di schizofrenia normativa che non tiene conto dell'evoluzione e della realtà dei fatti lo troviamo anche a proposito del ribasso dei listini dei farmaci. Tutti comprendiamo che sarebbe bello spendere poco o pochissimo per i farmaci che acquistiamo. Quindi, il fatto che la manovra finanziaria renda strutturali i tagli ai prezzi dei farmaci anche per gli anni a venire possiamo, ad una analisi superficiale, ritenerlo un fatto positivo. Ma se poi andiamo a comparare la crescita della spesa farmaceutica nel nostro Paese nell'ultimo quinquennio (1,7 per cento) con quella degli altri Paesi dell'UE (Germania 5,9 per cento, Austria 20,2 per cento, Regno Unito e Spagna oltre il 40 per cento), ben comprendiamo che cerchiamo la soluzione ad Est quando il problema viene da Ovest. Il problema si trova in chi gestisce la spesa sanitaria farmaceutica. Allora, cosa facciamo? Penalizziamo stabilmente i produttori dei farmaci! In questo modo sopprimiamo fìsicamente le nostre aziende e conseguentemente la ricerca nel campo della farmaceutica e della medicina, ma non intacchiamo l'inefficienza, o peggio, di chi gestisce gli acquisti e la distribuzione dei farmaci. Credo che l'esempio di questa legge finanziaria campeggerà a lungo nei testi di politica economica, magari confrontato con le strategie di Einaudi (e Menichella) del primissimo dopoguerra, le quali ultime fortunatamente hanno favorito il miracolo economico postbellico. Voglio ricordare - parlando di imposte, appunto - la via proposta da Einaudi che mi sembra, ieri come oggi, la più idonea ad essere perseguita: «L'ottima imposta «L'ottima imposta non è necessariamente alta o bassa; ed ottima può essere un'imposta del 20 per cento e preferibile a quella del 5 Ottima è quell'imposta data la quale, in un dato momento e luogo, si ottiene il miglior soddisfacimento dei bisogni pubblici compatibilmente con la produzione del più abbondante flusso di reddito nazionale. ottimo è quell'incremento di imposta il quale si adatta all'equilibrio economico preesistente e meno lo turba, con il minimo attrito, con il massimo rendimento per lo Stato e col massimo incremento del reddito privato. Ottima è l'imposta per la quale non diminuisce, ma cresce l'ammontare del reddito nazionale in confronto di quello che sarebbe stato senza di essa». Mi chiedo, se fosse presente e avesse analizzato la politica delle imposte di questo Governo e questa finanziaria, cosa penserebbe Luigi Einaudi. Naturalmente è un pensiero che voglio affidare soprattutto al ministro dell'economia Padoa-Schioppa. Credo superfluo ricordare le condizioni in cui Einaudi operò, in un Paese ad inflazione devastante, distrutto dalla guerra, sia nelle sue strutture pubbliche che in quelle dell'economia privata. In conclusione, le scelte scellerate che pervadono quasi tutta la legge finanziaria soggiacciono a delle ragioni anti-economiche, con una interpretazione della funzione del bilancio pubblico come strumento di attuazione di mere concezioni ideologiche dell'economia, totalmente estraneo all'economia liberale e concorrenziale. La rendita, come espressione economica del benefìcio della posizione e dell'oligarchia politica e finanziaria, è fotografia perfetta di una situazione statica e sopraffà il profìtto, come risultato delle componenti del conto economico, perenne confronto tra costi e ricavi, dinamica dell'efficienza e dell'evoluzione competitiva. Nel giudizio su questa finanziaria dovremmo saper scegliere tra importanti pareri: dell'Unione Europea, che plaude ed approva il rispetto dei parametri, sorda e cieca, o meglio disinteressata, all'economia vera e complessa, e le agenzie di *rating*, che valutano il sistema nel suo insieme e che si preoccupano tanto del bilancio e dell'efficienza dello Stato quanto quello del sistema produttivo, della sua competitività internazionale, delle capacità d'investimento e progettualità. La bocciatura che da queste ultime è giunta all'attuale manovra finanziaria esprime senza dubbio il giudizio più autentico, imparziale, concreto, a cui dobbiamo fare fede per quando sarà tempo, a breve, di invertire questa rotta.

Onorevoli colleghi, Governo e Parlamento sono stati impegnati negli ultimi sei mesi al varo di questa finanziaria, la quale è stata al centro della comunicazione mediatica per almeno gli ultimi tre mesi. Caricata forse di tante, troppe attese dopo cinque anni di crescita zero del Paese e di mancate riforme liberali, la manovra è stata accolta negativamente dal disorientamento dell'opinione pubblica e, in una certa misura, dalla stessa classe politica, incapace in parte, nella stessa maggioranza, di spiegarne le ragioni ed il senso, la cosiddetta *mission*. E così erano in tanti sabato 2 dicembre a sfilare per le vie di Roma contro le tasse. Ma le proteste fiscali a cavallo fra due legislature non chiamano mai in causa un solo Governo. Come Tremonti e Visco si contendono il merito del *boom* delle entrate e, dunque, dell'incremento della pressione fiscale nel 2006, così la rivolta contro le tasse non può che scaturire anche dalle leggi di bilancio della passata legislatura. Le finanziarie tra il 2002 e il 2005 ci hanno lasciato in eredità una crescita di due punti del rapporto fra spesa pubblica primaria e prodotto interno lordo, dal 42 al 44 Il Governo Berlusconi, in quegli anni solidamente al potere, ha obbligato tutti gli italiani, inconsapevolmente, a firmare una cambiale esigibile dal primo Governo che fosse fiscalmente responsabile. I DPEF della passata legislatura hanno applicato la strategia degli annunci, promettendo imminenti e consistenti sgravi IRPEF alle famiglie, tagli all'IRAP pagata dalle imprese e annunciando una lunga serie di misure spesso poi inattuate. È stata una consapevole strategia dell'illusione. Viene perciò legittimo chiedersi se Berlusconi, quando era alla guida del Governo, sapesse davvero cosa bisognava fare e, dato che dal palco di Roma non si è udita una sola parola di autocritica sulla gestione dei conti pubblici nella passata legislatura, l'interrogativo rimane e rimarrà attuale. Nella manovra economica proposta da questo Governo vi è finalmente una discontinuità importante rispetto alla legislatura appena iniziata. Si è cominciato a passare, ne siamo convinti, dalla politica degli annunci a quella dei fatti. il DPEF è consapevole del fatto che l'unico modo per risanare i conti pubblici risiede nell'abbassare il rapporto fra spesa pubblica e PIL e identifica le aree cruciali per interventi di contenimento della spesa. A differenza del suo predecessore, l'attuale Ministro dell'economia ha dato già prova che sotto la sua guida l'Italia onorerà i debiti, evitando di ricorrere a *una tantum* creative. Il ministro Padoa-Schioppa afferma oggi in una intervista: sono sereno, l'Italia ci capirà. Poiché è persona seria e ritengo creda nella politica dei fatti, egli ha fiducia che, passato lo tsunami mediatico-politico, questo Governo riconquisterà la fiducia degli italiani, perché finalmente si cominceranno a vedere i fatti. Molti dicono che non si vede la *mission* di questa manovra. Ebbene, dopo il passaggio al Senato, la *mission* è scritta nero su bianco all'articolo 1 della finanziaria, dove si dispone che le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 saranno destinate prioritariamente a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, ma, in quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale. Dunque, primo obiettivo: ridurre il nostro debito pubblico perché la sua dimensione, in assoluto e non solo in rapporto al PIL, ci rende molto vulnerabili al rischio di turbolenze sui mercati finanziari internazionali. Siamo nelle loro mani, nel senso che i nostri titoli di Stato sono detenuti oggi per più di metà da investitori esteri, molti dei quali istituzionali, non più dalle nostre famiglie, come era nel passato. Chi oggi propone di limitarsi a stabilizzare il debito ama probabilmente giocare alla roulette russa. adottare come strumento fondamentale la lotta all'evasione fiscale. Se è innegabile che l'obiettivo di riduzione del *deficit* viene raggiunto con un aumento delle entrate nette dello Stato, tuttavia, non tutte le entrate rappresentano un aumento di prelievo netto aggiuntivo sul settore privato. I proventi della lotta all'evasione fiscale, appunto, oltre a rispondere a un'ovvia esigenza di equità, non sono un prelievo aggiuntivo su cittadini e imprese che già adempiono al loro dovere fiscale e non hanno un effetto recessivo nel medio periodo, perché una riduzione dell'evasione fiscale comporta anche una riduzione delle distorsioni della concorrenza tra soggetti altrimenti uguali. Terzo obiettivo: la *mission*, puntare alla crescita e all'equità sociale. Abbandonato l'armamentario ideologico del passato, l'articolo 1 di questa finanziaria riconosce che la ricchezza, per essere distribuita, va prima prodotta. Il Governo, questa maggioranza, dimostrerà di voler e saper sostenere in questo Paese chi lavora e chi produce, l'Italia fatta anche dalle tante piccole e medie imprese che combattono sui mercati, che innovano, che non si arrendono. Questo è lo dico per inciso, anche un problema politico vero per la nostra maggioranza, quello di colmare la distanza con la parte più produttiva, vivace, dinamica della società italiana. Se dunque l'oggetto di un nuovo patto sociale è innanzi tutto lo sviluppo, la crescita, la produttività dei fattori, bisogna ultimare quanto prima il cammino di questa finanziaria per mettere subito mano alle riforme (liberalizzazioni, semplificazione amministrativa, riforma della pubblica amministrazione, infrastrutture materiali ed immateriali, federalismo). Un piccolo accenno sul federalismo. In questa finanziaria sono state accolte due proposte, ai commi 143 e 704 del maxiemendamento, che costituiscono a mio avviso delle innovazioni fondamentali. Al comma 143 si stabilisce che l'addizionale comunale all'IRPEF sarà versata dal periodo di imposta 2007 direttamente ai Comuni. È un'innovazione in senso autenticamente federalista, possibile a Costituzione vigente. Al comma 704 viene stabilita finalmente una misura premiale per gli enti locali che rispetteranno il Patto di stabilità nel 2006.

sarà distribuito esclusivamente ai Comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2006. L'articolo 1 dice anche altro, cioè che bisognerà mettere mano alla riduzione della pressione fiscale, perché sappiamo che una politica incentrata sull'aumento delle tasse nel medio periodo blocca la crescita e genera instabilità politica. Una prima scadenza, lo dice sempre l'articolo 1, sarà sul punto il prossimo 30 settembre, quando si dovrà verificare seriamente la possibilità di ridurre la pressione fiscale che, dal 2005 al 2007, è previsto un aumento di oltre due punti. Ma insieme alla crescita e allo sviluppo, a noi sta a cuore l'obiettivo fondamentale dell'equità sociale. La stella polare della nostra politica è infatti l'eguaglianza, non l'egualitarismo. Una politica egualitaria è caratterizzata, secondo la nota distinzione di Bobbio, dalla tendenza a rimuovere gli ostacoli, per riprendere l'espressione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, quegli ostacoli che rendono gli uomini e le donne meno uguali. uguali. Una politica riformista, infatti, non si arrende alle diseguaglianze, non le accetta come un fatto ineluttabile, ma pone in essere ogni iniziativa volta a porre gli uomini e le donne sulla stessa linea di partenza nella competizione della vita.

vista la veemente reazione dell'opinione pubblica a una finanziaria che è stata fatta passare come quella che aumenta la spesa e le tasse proprio da chi lo ha fatto già con successo per i cinque anni precedenti. forse non siamo riusciti a comunicarlo perché, dopo tanti anni di politica degli annunci, gli italiani sono disincantati, non credono più ai proclami della politica e forse anche perché questo Paese è un po' contraddittorio. Gli italiani sono affetti, scriveva scriveva ieri Ilvo Diamanti su «la Repubblica» da strabismo etico: vogliono che i servizi sociali restino in mano al pubblico, ma ne sono insoddisfatti; si rendono conto che bisogna riformare le pensioni, ma si oppongono a una riforma che allunghi l'età pensionabile; sono d'accordo sulle liberalizzazioni, ma non per la propria categoria, per il proprio ordine professionale; non vogliono vogliono aumenti delle tasse, ma non accettano neppure riduzioni della spesa per i servizi; chiedono legalità, ma sono indulgenti verso i comportamenti illeciti in ambito sociale ed economico. Gli italiani che oggi protestano forse pensavano che bastasse cambiare la guida del Paese perché le cose andassero meglio; sono delusi e diffidenti, non solo da oggi, verso la classe politica e forse ne hanno ben ragione, perché la classe politica è stata prigioniera, in tanti anni, del consenso ed incapace di fare le riforme nell'interesse generale quando questo costa in termini di consenso. Urge dunque passare dalla politica degli *slogan* alla politica dei fatti. Se il centro‑sinistra vuole continuare a governare, se ambisce a farlo per almeno due legislature, il tempo minimo per completare le riforme strutturali necessarie a far ripartire il Paese, deve davvero mettersi a fare, e al più presto, le cose che sappiamo di dover fare, quelle annunciate nel DPEF con coraggio e lucidità, come si è fatto del resto con la scelta di privatizzare Alitalia, bloccando il drenaggio di denaro pubblico e lasciando al mercato la decisione sulle alleanze. Questo è un esempio concreto, un fatto, del cambiamento di rotta rispetto al passato: solo così si convincerà il Paese. Il Paese, signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è già oltre questa finanziaria. Mettiamoci, dunque, subito al lavoro per fare le riforme, non ultima quella della sessione di bilancio, perché il Paese non può premettersi più di investire così tanto tempo in una sola legge, lasciando che su una partita così importante prevalga, come è prevalsa, la logica dell'appartenenza e della contrapposizione politica, anziché quella della responsabilità istituzionale nell'interesse generale del Paese. Auguro, dunque, buon lavoro al Governo, auspicando sin dall'inizio del prossimo anno un confronto e una collaborazione ancora più continua e proficua tra esso e il Parlamento nell'interesse generale del Paese. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, gli annali della storia nazionale annovereranno l'intera vicenda di questa legge finanziaria di questa legge finanziaria come il punto culminante della crisi politica istituzionale che ha colpito l'Italia e che si trascina ormai da alcuni anni. Il mio non è un giudizio apodittico di parte, ma è la constatazione del punto in basso al quale è pervenuta questa vicenda. In altre epoche la centralità del Parlamento, il rispetto rigoroso delle regole procedurali era il punto fermo delle posizioni politiche di opposizione, ma era, al tempo stesso, il limite al quale si attenevano rigorosamente le forze di Governo. discutibile introduzione della legge finanziaria fu determinata, negli anni Settanta, dalla precisa istanza di inchiodare il Governo a scelte di finanza pubblica controllate e fermamente determinate dal Parlamento, in coerenza con l'essenza stessa del Parlamento, che sorge, nella sua prima manifestazione storica, per controllare le tasse stabilite dal re e l'uso che egli stesso ne avrebbe fatto. Orbene, il Governo si è prestato a portare, nella forma del *diktat* - non si può definire diversamente - implicato dalla questione di fiducia, un disegno di legge finanziaria inqualificabile sotto l'aspetto procedurale, ma anche molto discutibile, e per me inqualificabile, sotto il profilo sostanziale. Mi sembra quasi singolare - l'ho sentito da alcuni colleghi della maggioranza ricordare che la legge finanziaria dovrebbe essere composta da pochi articoli. È vero, è anche invalso in altro tempo una procedura diversa, ma mai si era arrivati al punto odierno, in cui il Parlamento (il Senato, nel nostro caso) deve esaminare un testo di commi, neppure di articoli, che dovrà votare con il tasto rosso o con il tasto verde. È innanzitutto sotto questo aspetto che essa va fermamente contestata, perché la procedura parlamentare è una condizione essenziale della regola democratica. Così si ha soltanto uno svuotamento totale del Parlamento, ridotto a ratificare o a disapprovare. Nel merito poi - ed è stato ampiamente motivato da molti interventi - abbiamo

dà il risultato di una sopravvenienza molto forte, si verifica un prelievo fiscale in misura non giustificata da razionali fini ed obiettivi. Il risanamento non è collocato in una prospettiva, anche temporale, che dovrebbe aggredire o almeno ridurre lo *stock* del debito pubblico. La norma contenuta nel primo comma di questa legge finanziaria - lo sanno tutti, onorevoli senatori - è soltanto una norma *slogan*, una norma manifesto, che non avrà alcuna concreta conseguenza e alcun concreto seguito. Anzi, c'è addirittura uno scarto, un salto logico di proporzioni sconvolgenti, tra questa legge finanziaria e il DPEF, pur criticabile, come lo è stato da parte nostra; ma in prospettiva positiva il DPEF accennava e disegnava una strategia per la finanza pubblica e per l'economia del Paese. Adesso è stato compiuto un salto all'indietro, un salto nel buio. Le risorse prelevate che si cumulano con le sopravvenienze del gettito tributario - effetto di una ripresa economica indotta dalla generale ripresa registrata quest'anno dall'area europea e, segnatamente, dalla locomotiva tedesca non vengono utilizzate minimamente per finalità che possano essere il segno di un progetto per il Paese. Qualcuno

Alla presentazione della legge finanziaria con il Ministro dell'economia alcuni suoi colleghi avevano cantato il ritornello:equità risanamento e sviluppo.

troverete che i ricchi (con la «r» maiuscola) hanno portato, ciascuno di loro, un pacco dono più grande di quanto si possa immaginare. E, per somma ironia, il beneficio che è stato loro elargito non ha neppure assunto la forma di un incentivo finalizzato a una trasformazione dell'apparato produttivo, a una crescita delle strutture dell'industria italiana, a una promozione reale e concreta della ricerca e della ricerca applicata. Il beneficio è soltanto nella forma del sostegno della rendita: sarebbe bene che chi, qualche tempo fa, ha lanciato l'anatema contro le rendite, consideri alcune disposizioni erogatorie (e non sono a partire da quella rottamazione, reintrodotta dopo gli anni Ottanta, e che in quegli anni fu una droga per l'industria automobilistica; per non parlare poi di tanti altri pacchi dono.

il Governo, ancor prima del Parlamento, ad avanzare uno straccio di proposta di politica energetica, quando sappiamo tutti che la vera strozzatura che grava sull'economia del Paese,

per i consumatori, ma soprattutto per l'apparato industriale. La revisione delle aliquote, avanzata come mezzo di lotta all'evasione, come tutta la batteria delle misure fiscali, ha avuto soltanto un obiettivo: colpire i ceti medi,

come colpevole ed è vittimizzato. Facendo ciò, si compie un errore di strategia sociale, ancor prima che politica, come se fosse possibile nell'Italia del ventunesimo secolo immaginare di regredire alle estreme categorie del capitale da una parte e, dall'altra, del lavoro dipendente. Sarebbe, invece,

di lavoro autonomo e creativo che fanno la sostanza di un rinascimento che, quando conviene, viene glorificato. Sulla politica fiscale si insiste sull'opposto della scelta che altre Nazioni hanno effettuato in questi anni, dove la riduzione dei carichi fiscali ha avuto un effetto incentivo per lo sviluppo economico e per la stessa lotta all'evasione. Era questa la linea su cui bisognava insistere, semmai temperandola - come è stato sempre indicato nelle proposizioni politiche dell'UDC dell'UDC - soltanto col privilegio da accordare alla famiglia in quanto soggetto di insieme, complessivo, in un'ottica che deve ricollegare sempre la politica fiscale ad una politica sociale che sia fondata sulla tutela e sulla promozione della famiglia, come ha mostrato di saper fare negli anni recenti anche la Francia.

Il Governo in questa manovra finanziaria non ha dato seguito concreto ad un'indicazione, pur contenuta nel DPEF: iniziare un percorso di riduzione dello *stock* del debito pubblico. Anzi, per tutti coloro che hanno fatto fortuna politica gridando allo scandalo del debito pubblico agli inizi del 2000, devo ricordare che nel 1993 il debito pubblico era il 115 per cento del PIL, nel 1995 il 121,20 2005 il 106,60 per cento. Non credo che possa essere diverso nel 2006 e neppure nel 2007, ammesso che la spesa pubblica non continui a crescere, così come si contesta al Governo precedente Onorevoli senatori nonostante i prelievi fiscali di portata eccezionale come quelli del Governo Amato del 1992 e quelli di Prodi oggi lo *stock* del debito pubblico rimane intatto. Ma, per contro, non ci sono più i gioielli di famiglia, sono stati tutti dati via. Le privatizzazioni, da chiunque portate avanti (non ci vuole molto né a farne l'elenco, né a indicarle), hanno dato quei dieci punti che hanno fatto scendere il monte del debito pubblico al livello attuale. Ed ora? Il Governo Prodi avrebbe potuto imboccare il sentiero, stretto e lungo, che occorrerà percorrere se si vuole lavorare sul costo del debito, che ascende a 76 miliardi di euro (dicasi qualcosa come 140.000-150.000 miliardi delle vecchie lire) e che rappresenta una condizione di ostaggio in cui viene tenuta la finanza pubblica. Anzi perché non dirlo - alla sovranità dello Stato è subentrata la sovranità dei mercati e il *rating* delle agenzie ormai è più importante del voto del popolo. Una forza politica, che viene dalla storia della rappresentanza del lavoro e che ha ritenuto le ragioni di classe un fondamento della propria missione ideale e della propria proposta politica,

Accogliere questa sfida è qualificare la propria posizione riformista. Questo non è avvenuto. Guardando la legge finanziaria, si si assiste ad una pioggia di finanziamenti, qualcuno dei quali è anche condivisibile, ma trattasi comunque di finanziamenti a pioggia (come si diceva una volta), che alimentano soltanto l'area della spesa di taluni Ministeri in funzione di alcuni obiettivi.

del metano nella Val Padana un progetto di unificazione del Paese ed in quel contesto non un siciliano o un meridionale, ma uno proveniente da Varese, senatori della Lega, Lega, seppe proporre a De Gasperi l'istituzione dell'intervento straordinario. Della questione meridionale, in questa legge finanziaria, non si trova traccia in positivo.

un trattamento che ha subito la sua comparazione nell'articolo successivo. Orbene, il Governo con questa legge finanziaria si è voluto dare la zappa sui piedi. Non ci si lamenti delle manifestazioni in piazza! Nel Paese crescerà un dissenso profondo ed inarrestabile nei confronti di un Governo che ha fatto la scelta peggiore, quella di mantenere la sua maggioranza purchessia.

Da più parti, oramai, si ritiene che le procedure di costruzione ed approvazione della legge finanziaria debbano essere profondamente modificate, per porre fine alla deformazione che la finanziaria ha subito con il passare degli anni. Una legge finanziaria non può cambiare o cancellare gli effetti prodotti dai Governi precedenti, non può dare risposte tali da modificare radicalmente le condizioni sociali stratificate nel tempo; può però dare il segno del cambio di marcia, della scrittura di una nuova pagina in cui il tema dell'equità e della giustizia sociale assumono la centralità nell'intervento. Non si può però dare un giudizio sull'efficacia di questa finanziaria senza partire dalle condizioni economiche e sociali ereditate dai Governi precedenti. Un'eredità pesante, fatta di profonde lacerazioni sociali e territoriali, di precarietà e insicurezza, di povertà di settori sempre più estesi della nostra società e di nicchie di privilegi e di accumulazione della ricchezza intollerabili. La finanziaria nasce dunque con l'obiettivo di intervenire sui tre pilastri del risanamento dei conti pubblici disastrati, dell'equità e dello sviluppo. È con questo spirito che il nostro partito ha agito in questi mesi, intervenendo per modificare il testo della finanziaria giunto in Parlamento. Ci siamo posti alcuni obiettivi, che in larga parte vengono recepiti nel testo del maxiemendamento. Sarebbe sbagliato oggi far prevalere nelle nostre analisi e nella comunicazione esterna un senso di delusione per alcuni errori e per alcune scelte che non condividiamo, che sono state inserite nelle ultime ore senza il dovuto confronto con la maggioranza. Tali errori andranno immediatamente corretti, per dare un senso compiuto al lavoro che in queste settimane le senatrici e i senatori dell'Unione hanno prodotto per migliorare il testo della finanziaria. Ci sono positivi elementi di discontinuità, rispetto alle manovre del centro-destra, a partire dalla riforma dell'aliquota IRPEF e del nuovo regime di detrazione e di assegni familiari, che avviano una redistribuzione delle risorse verso le fasce più deboli e di reddito più basso. Così come, dopo gli anni dei condoni fiscali, si avvia una lotta seria all'elusione e all'evasione fiscale che sta cominciando a produrre i primi risultati. Come non vedere l'attenzione che viene posta al tema del lavoro e della lotta alla precarietà con misure importanti in tema di diritti lavoratori precari, dalle maternità a rischio alle condizioni di malattia, come spiegato ieri dal senatore Zuccherini. Siesprime, ad esempio, forte soddisfazione per il recepimento nel maxiemendamento della nostra proposta di dare un segnale chiaro e visibile della volontà di una lotta senza quartiere agli incidenti sul lavoro e alla tragedia delle morti bianche, quattro al giorno, di cui il nostro Paese detiene un triste primato. Assumere 300 nuovi ispettori del lavoro va in questa direzione. Ricordo, senza polemica, ai colleghi del centro-destrache nei cinque anni precedenti in quest'Aula è stato sempre presentato questo emendamento senza che venisse mai una risposta. Non voglio tornare sugli aspetti positivi su cui si sono già intrattenuti i miei colleghi, tra cui la senatrice Capelli, sugli importanti risultati ottenuti nel mondo della scuola, con la stabilizzazione dei precari, o sulla sanità con l'abolizione dei *ticket*. evidenziano molti tratti positivi che danno il senso del cambiamento e della volontà di agire nello spirito dell'equità, della giustizia e dell'attenzione sulle tematiche ambientali. Restano alcune ombre, alcune indecisioni che vanno rapidamente superate. Nel poco tempo che mi resta a disposizione voglio affrontare il nodo delle politiche energetiche e dell'errore di scrittura nel testo sul tema del CIP 6. Il CIP 6 non è un'impuntatura della sinistra radicale o di una parte della maggioranza, ma una delle maggiori truffe legalizzate della storia del nostro Paese che dal 1992 continua a regalare miliardi di euro, sottratti dalle bollette pagate dai cittadini, ai grandi gruppi industriali, ai petrolieri, alle *lobbies* degli inceneritori che hanno anche qui dentro molti portavoce. Voglio rimanere alle comunicazioni del Governo secondo cui si è trattato di un mero errore di scrittura. dunque che questo Governo vuole cancellare lo scandalo dei CIP 6. Saremo tutti più tranquilli - mi rivolgo ai rappresentanti del Governo presenti - se l'Esecutivo ci dicesse come intende correggere l'errore. Vorrei solo rispondere al ministro Bersani che non si può discutere del pacchetto energia e del disegno di legge presentato in Senato senza prima aver risolto questo problema. Aspettiamo dunque un segnale immediato già questa sera, prima del voto, sulla procedura che il Governo intende adottare per superare questo errore. Penso che, nei prossimi mesi, nell'Unione si debba aprire una discussione seria e vera sulle grandi questioni che riguardano gli interessi dei cittadini di questo Paese, senza disperdersi nei vicoli ciechi suggeriti dalla Confindustria o dai settori economici più influenti. Non mi voglio attardare sulla definizione semantica più corretta per definire l'esigenza di cambiamento dell'agire politico del Governo Prodi, fase due o cambio di passo che dir si voglia. Lo slancio che si deve dare è quello delle riforme, riforme vere, che devono liberare uno spazio di progresso sociale per migliorare le condizioni di chi oggi sta peggio nel nostro Paese. Le critiche e i limiti della finanziaria devono rappresentare lo stimolo per costruire il consenso attraverso una maggiore partecipazione democratica ai processi decisionali. Bisogna continuare con più coraggio sulla strada dell'equità e dello sviluppo. Ci attendono mesi in cui bisogna affrontare nodi importanti e l'unico modo per evitare incomprensioni con il Paese è il rispetto del programma, punto di riferimento sul quale abbiamo abbiamo ottenuto il consenso e vinto le elezioni. Diamo un'anima alla nostra azione e teniamo alta la speranza di futuro per le nuove generazioni. il Senato si accinge tra qualche ora ad esprimere il suo voto su una legge finanziaria e di bilancio che risulta già essere stata bocciata nel Paese e dal Paese. Mai, come in questa occasione, un atto legislativo del Parlamento italiano aveva suscitato l'interesse mediatico e il risentimento della piazza. Mai gli italiani tutti, di ogni ceto sociale ed età, si sono sentiti coinvolti e toccati nel profondo ed hanno reagito a quel senso di incertezza ed instabilità che, al contrario di quello che proclama il presidente Prodi, non può non dilagare e dilaniare tutti gli onesti lavoratori italiani. È il colpo di grazia dopo una serie di provvedimenti «bandiera», fatti o annunciati, che presentano agli italiani un modello di società che il centro-destra non può non combattere e avversare con forza. In pochi mesi ci si è preoccupati di aumentare la dose consumabile di *cannabis*, di fare un indulto che non ha precedenti per dimensioni, di regolarizzare nella realtà dei fatti 350.000 immigrati clandestini con il provvedimento sui flussi ed ora si parla di Pacs e di eutanasia. Una rivoluzione copernicana non solo rispetto al Governo Berlusconi, ma anche rispetto a quel modello «ordinato» di società che la Democrazia Cristiana per decenni dal dopoguerra aveva difeso e che oggi alcuni eredi della stessa DC contribuiscono a destabilizzare e cancellare. La stessa finanziaria nasconde un progetto preciso e di lungo termine di «riforma» della società e dei suoi assetti economici e può essere compresa e letta solo insieme al decreto Bersani-Visco e al decreto fiscale. Così come questi due provvedimenti avevano colpito i ceti medi, ma soprattutto i corpi intermedi della società italiana, anche questa finanziaria, nata marcatamente ideologizzata e poi disordinatamente rivisitata, muove dalla stessa idea che là dove c'è o si sa creare ricchezza, e questo è più grave, si deve colpire inopinatamente. Vale la pena di ricordare tutte le difficoltà politiche di questa finanziaria. Innanzi tutto, il grande *bluff* dei dati: 37 miliardi di euro di maggiori entrate nel 2006 grazie al precedente Governo minimizzati da Visco. E poi la grande abbuffata: una manovra da 35 miliardi di euro circa, come nemmeno l'Unione Europea richiedeva. Lo sconcerto politico di tutti i Ministri sul documento del ministro tecnico Padoa-chioppa, i quali corrono ad emendare ed emendare ancora. Il giudizio della finanza internazionale e quello dell'Unione Europea. Le minacce di non voto dei senatori a vita. Le centinaia di manifestazioni di piazza e gli scioperi. L'ostruzionismo della maggioranza alla maggioranza, con le migliaia di emendamenti dei deputati e dei senatori di centro-sinistra. La non conclusione dei lavori delle Commissioni bilancio. Ed infine, i voti di fiducia. L'evidenza di questa finanziaria è un Consiglio dei Ministri in lotta intestina e un Governo che si beffa dei suoi Gruppi parlamentari. Ma il fatto più grave più grave è che, facendo la maggioranza opposizione a se stessa e al suo interno, questa vuole impedire alla vera opposizione parlamentare di esercitare il suo ruolo, così come il Governo continua ad esautorare il Parlamento delle sue prerogative. Anche gli agricoltori, come tutti gli imprenditori pesantemente irrisi e colpiti, pagheranno il loro pegno, non solo quello della «confisca del TFR». È noto che le misure che riguardano il cuneo fiscale incidono in maniera assai lieve sul settore agricolo. Ci aspettavamo e avevano chiesto misure strutturali per l'agricoltura italiana. Se non si affronta il nodo del costo del lavoro in agricoltura (con riduzioni delle aliquote INAIL, ad esempio) non ci sarà mai l'emersione del nero e del lavoro extracomunitario irregolare. Nessuna misura per il riaccorpamento fondiario, che è un problema strutturale e vecchio, ma ora assolutamente urgente. E poi perché dimenticare sempre - salvo salvo poi rimediare in *corner* e in maniera assolutamente parziale - che la terra, come il lavoro, è in agricoltura il principale fattore della produzione e questo vale per gli imprenditori singoli come per le società, per le piccole e per le grandi aziende, e che ogni tre generazioni non si può riacquistare con la tassa di successione e parlo con un'allitterazione voluta - la propria proprietà. Pesante sarà il contributo degli agricoltori a questa finanziaria anche con la deruralizzazione dei fabbricati. Poco o niente contiene sul fronte della semplificazione amministrativa di cui l'agricoltura ha tanto bisogno, o per favorire l'accesso al credito delle aziende agricole che mostrano sofferenza di liquidità a causa di annate pregresse che hanno registrato calamità, emergenze fitosanitarie e un calo vertiginoso dei prezzi. Anche sul piano irriguo, sul quale l'opposizione si è battuta in Commissione, si poteva fare di più. In generale, pensiamo che questa finanziaria si preoccupi più dell'agricoltura di nicchia che di difendere dalle sfide del mercato e della competitività la nostra grande agricoltura tradizionale, che è l'identità italiana. Ora aspettiamo con terrore la seconda finanziaria, cioè le maggiori imposte (ICI, IRPEF, accise e quant'altro) che le Regioni e i Comuni saranno legittimati a imporre proprio grazie a questa finanziaria e alla scelta politica di operare minori trasferimenti agli enti locali. Concludo queste breve riflessioni con una considerazione che fa ancora riferimento a quella grande rivoluzione culturale che la sinistra, non solo in Italia, sta operando, travolgendo valori, tradizioni e identità per approdare non si sa bene dove e a che cosa. Se gli aeroporti inglesi, dopo aver montato gli alberi di Natale, li smontano, se negli Stati Uniti e nelle comunità anglosassoni sta scomparendo la parola *Christmas* dai biglietti di auguri e in Italia si vendono meno Presepi, speriamo almeno che la superstite Befana porti al presidente Prodi e ai suoi Ministri solo tanto carbone.

(prima il decreto‑legge fiscale, poi la legge finanziaria), la prima reazione è stata di sconcerto. Come mai un Governo del rigore, un Ministro dell'economia e delle finanze che ha fatto del rigore la cifra di un'esistenza producono, già all'ingresso, una finanziaria di 213 commi e un decreto-legge di 60 commi? La più lunga delle finanziarie che io ricordi in oltre undici anni, già all'ingresso. Com'è possibile? È ben noto che, se una finanziaria è così corposa sin dal suo inizio, ha due difetti: fa emergere evidentemente la confusione di chi la produce ed invita, durante il cammino parlamentare, a produrre tanti altri commi ed articoli. Eravamo facili profeti. Siamo giunti a 1365 commi, ai quali dobbiamo aggiungere quelli del decreto fiscale. Una bella cifra, non c'è che dire. Se foste arrivati a 2600, avremmo avuto la storia dell'umanità occidentale. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Speriamo che l'anno prossimo riusciate a fare questo, così potremo portare la vostra finanziaria per diseducare i bambini alla scuola. Ma come mai ciò è accaduto? È facile. Pensavate di farla franca perché, con una grancassa con una grancassa mediatica, avevate detto che il precedente Governo aveva lasciato un debito alle stelle e fuori controllo, un *deficit* fuori da ogni parametro europeo, una crescita bassissima e una dissennata politica fiscale. Se questo era il passato, se così grave era la situazione della Nazione (si parlava di eclissi e di declino immediato), dunque voi potevate far tutto, perché avevate il grande onere, il grave peso di dover risollevare la la situazione politica ed economica di questa Nazione. Ed allora subito vi date da fare e producete il decreto Visco-Bersani, con il quale cominciate, sul piano della politica fiscale, a creare un clima (che tutti i cittadini conoscono) di assoluta vessatorietà ed inconcludenza, come dirò. Le misure vessatorie già fanno male alla gente; quando sono vessatorie ed inefficaci, la irritano. È questa la ragione per cui siete sistematicamente fischiati: in maniera organizzata, che sarebbe un merito di chi fischia, o disorganizzata, se spontanea, ed è altrettanto un merito di chi si sente dalla vostra politica economica ingiustamente colpito. Non colpito; ingiustamente colpito. Nel corso della finanziaria siete smentiti clamorosamente: vi trovate infatti di fronte ad un aumento senza precedenti delle entrate fiscali. entrate fiscali. Signor Ministro, lei non ha avuto la cortesia di venire durante i lavori della Commissione bilancio; la pregherei, il prossimo anno, augurandole di restare, di essere un po' più solerte. Nella Commissione bilancio del Senato si discute con molto approfondimento ed attenzione. La sua presenza ci avrebbe rincuorati ed avrebbe portato un grande contributo; la sua assenza

in un contesto di riduzione della pressione fiscale. Dunque, era evidentemente vero che la nostra politica, riducendo le aliquote, quindi il peso su ciascun cittadino, aveva favorito l'emersione di una più larga base imponibile e dunque indotto un circolo virtuoso nel meccanismo fiscale. Cosicché i cittadini, sentendo in misura per lo meno parzialmente più giusta le imposte, le pagano. Niente a che fare - non mi soffermo molto - con le questioni di inizio finanziaria, che per fortuna non sono state ripetute, sui meriti di questo Governo. Lo sanno tutti che non c'entra niente questo Governo, perché si sta parlando di tasse che vengono dalle politiche precedenti. Vedremo l'anno prossimo i frutti della vostra legge finanziaria. Se fossimo utilitaristici, saremmo contenti visti gli scontenti, ma siamo persone che hanno governato l'Italia e puntano a governarla ancora: per questo siamo responsabili e non siamo contenti per il Paese. Questo è il quadro totalmente modificato che vi siete trovati di fronte e che non avete avuto il coraggio di modificare, anche se l'opposizione ve lo ha chiesto in più sedi durante tutto l'*iter* parlamentare della manovra e vi siete intestarditi.

la tassazione sulle locazioni, come avevamo proposto, ripromettendovi di provarci l'anno prossimo, lo spero per il Paese, ma io non ne sono molto convinto. A cosa si è ridotta nelle grandi cifre la vostra

i presunti proventi del TFR come possibile finanziamento delle infrastrutture. Consentitemi una battuta, forse un po' banale: speriamo che non capiti, ma ove mai il TFR sia stato

senza considerare comunque che il TFR, vivaddio, non sono soldi dello Stato, rimangono soldi dei lavoratori: si tratta di un vero e proprio esproprio. Ho già detto più volte che, se sotto il profilo delle leggi di contabilità pubblica questa è una manovra legittima, a mio avviso, sotto il profilo della politica economica di lungo periodo, essa è largamente azzardata e un tantino vessatoria nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sembra strano che a ricordarsi degli operai di Mirafiori

della linea economica che avete scelto, oltre che su un profilo una tantinello più basso, cioè sul piano della necessità di tenere unita la vostra coalizione, dando una qualche spruzzatina di sale e pepe a ciascuno degli innumerevoli Gruppi che compongono la vostra maggioranza. Vi devo ringraziare, questo sì, per la grande chiarezza, perché affianco ad ogni comma del

sul piano degli obiettivi strategici, non avete più avuto la bussola. Allora, l'unico modo di tenere insieme questa maggioranza era il collante di oltre

stanno a cuore l'Italia, la nostra gente, la nostra Nazione. Per questo, Signor Presidente, voteremo convintamente contro questa finanziaria, che sarà facilmente definibile la peggiore degli ultimi anni e, forse, della Repubblica Italiana.

Signor Presidente, interverrò in generale sulla legge finanziaria, ma prima di affrontarla nei suoi termini complessivi, credo di dover, in modo preliminare, riferire all'Aula la mia opinione sulla questione relativa alla norma contenuta nella legge finanziaria che si occupa di decorrenza dei termini dei giudizi davanti alla magistratura contabile. Nell'istruttoria in Commissione e in quella della maggioranza la norma era stata scartata, quindi considero la sua presenza nel testo finale frutto esclusivamente della concitazione con la quale la legge finanziaria viene

che, soltanto tre giorni fa, nell'Aula del Senato è stata accolta con un applauso unanime la denuncia del senatore Morando, il quale, visto il quadro normativo-regolamentare di cui disponiamo, ci ha ripetuto per l'ennesima volta

Ma c'è anche un problema di merito. E nel merito oggi posso solo dire che, come tutti i senatori dell'Ulivo, rispetto l'allarme della Corte dei conti e ne tengo talmente conto da chiedere anch'io al Governo di correggere il testo. Per completezza, che la versione originale dell'emendamento, che ha ispirato la norma poi contenuta nella finanziaria, aveva una formulazione diversa e prevedeva un secondo comma che avrebbe meglio definito e meglio regolamentato Adesso permettetemi di parlare più in generale sulla legge finanziaria. Permettetemi anche, in primo luogo, di ringraziare i senatori, di maggioranza e di opposizione, che vi hanno lavorato in Commissione e che ci hanno consegnato

che tra poco il Senato approverà e alla quale darò il mio voto con convinzione Ogni anno in Parlamento e fuori del Parlamento assistiamo a uno sportsingolare: la ricerca ossessiva di cosa c'è di sbagliato nella legge finanziaria, di cosa manca, di quali sono le sue contraddizioni. Dico subito che, date le regole del gioco, è uno sportfacile: che, date le regole del gioco, è uno sportfacile: in testi tanto complessi, redatti in condizioni materiali così improprie, è pressoché impossibile non cadere in errore. Ho evitato la demolizione sistematica delle leggi finanziarie anche quando, nella passata legislatura, ero all'opposizione e ritenevo di avere validissimi argomenti per farlo. Tanto più me ne sottraggo oggi che sostengo il Governo Prodi e ritengo, in piena coscienza, che la manovra che stiamo esaminando sia nelle sue linee portanti quella che oggi serve all'Italia. Badate bene, lo dico all'opposizione, non sto dicendo che non vi siano norme che potevano essere scritte meglio o che non vi siano norme mancanti. Sto solo dicendo che ogni legge finanziaria deve essere giudicata partendo dalla consapevolezza dei problemi del Paese, sapendo che l'elaborazione trova fondamento in norme legislative e regolamentari assolutamente inadeguate, conoscendo qual è la disponibilità delle risorse, tenendo presente che un giudizio politico corretto sul contenuto di ogni legge finanziaria non può prescindere dal considerarla inserita nell'attività complessiva del Governo, quindi in quanto il Governo ha fatto prima e nei programmi per il futuro e, per quel che riguarda questo Governo, nei programmi di riforma che il Governo ha annunciato e che giustamente ha escluso dalla legge finanziaria ed ha lasciato ad una discussione e ad una elaborazione successiva. È È sulla base di queste considerazioni di fondo, oltre che per il suo specifico valore, che esprimo un giudizio positivo sulla manovra e sento di poter dire che questa è la manovra che serve oggi al nostro Paese. Permettetemi di essere sintetico e di confidare che voi conosciate gli elementi che caratterizzano questo momento della storia d'Italia. Confido che il Parlamento abbia ben chiaro le caratteristiche del nostro Paese, perché con molta franchezza che sia al Governo che a noi parlamentari della maggioranza può essere addebitato un eccesso di prudenza in questo inizio di legislatura, forse addirittura una reticenza nel non aver voluto, nel non aver saputo indicare in modo chiaro e con la forza necessaria quali siano i fondamentali reali della nostra condizione economica, quanto profonde siano le crisi delle istituzioni pubbliche nazionali e regionali, in quali difficoltà si dibatta dibatta il nostro sistema produttivo e quali siano le debolezze del nostro Stato sociale. In una parola, credo - lo dico al Ministro dell'economia che né in campagna elettorale, né dopo, il centro sinistra non ha mai saputo dire con chiarezza e con la forza necessaria quale danno alla finanza pubblica e alle nostre istituzioni è stato procurato dai cinque anni di Governo che ci hanno preceduto. La legge finanziaria che stiamo esaminando vale circa 35 miliardi ed è una manovra quantitativamente gigantesca; è la seconda nella storia della Repubblica per dimensioni. Un terzo circa di questa manovra è stato utilizzato per riportare i nostri conti pubblici entro i parametri concordati con l'Unione Europea. Non mi sembra poco visto che, a fronte di un vincolo del 3 per cento, quest'anno il rapporto tra *deficit* e PIL raggiungerà la percentuale stratosferica tra il 6 ed il 5 per cento e che, proprio grazie a questa manovra, nel 2007 rientreremo finalmente nel limite del 3 per cento prescritto dal Patto di stabilità e di crescita. Un'altra parte delle risorse è stata impiegata per soddisfare impegni già assunti, le cosiddette spese obbligatorie. A cominciare - mi piace ricordarlo - dagli investimenti nei grandi servizi pubblici essenziali quali l'ANAS e le Ferrovie dello Stato, ambedue portate dal Governo di centro-destra a condizioni prefallimentari. Uso l'espressione «prefallimentare» in senso tecnico non in senso figurato. Un'altra parte della manovra, infine, è stata posta a servizio dello sviluppo. Qualcuno dell'opposizione ha sostenuto che la finanziaria poteva essere più leggera. Cosa si voleva dire? dire? Se qualcuno chiedendo una finanziaria più «leggera» ha voluto dire che non era necessario investire nello sviluppo del Paese, gli consiglierei di riflettere meglio prima di parlare. Nel 2001 l'Italia era al 24° posto nella classifica della competitività globale, mentre a fine 2005 era finita al 47° posto e non credo che la responsabilità di questa catastrofe possa essere addebitata al centro-sinistra. C'è un dato reale da cui dobbiamo partire se vogliamo capire la natura profonda della crisi. Questo dato è costituito dall'intreccio che lega il nostro mostruoso debito pubblico gli abnormi interessi che ogni anno siamo costretti a pagare per onorarlo; lo lega con la debolezza delle politiche economiche che proprio la ristrettezza delle risorse ci permette di promuovere. Di qui l'importanza sia del risanamento, che di una politica per lo sviluppo, perché l'uno senza l'altra sono impossibili. A proposito di sviluppo, faccio solo rilevare la straordinaria portata della nuova normativa fiscale, che porterà ad un incremento del gettito senza inasprire i contributi e che introduce il principio fondamentale, e per l'Italia rivoluzionario, che i risultati della lotta all'evasione (che già si preannuncia particolarmente efficace) dovranno produrre una corrispondente riduzione del peso fiscale. Faccio anche rilevare all'Aula l'attenzione al rilancio della politica industriale e delle competitività delle imprese (in primo luogo, delle piccole imprese) attraverso la riduzione del costo del lavoro, il credito d'imposta per le spese di ricerca, la revisione delle regole sugli studi di settore, le agevolazioni per gli apprendisti e così via. Egualmente faccio rilevare - l'ho già citata prima - l'inversione della politica per le infrastrutture (mi riferisco nuovamente all'ANAS e alle FS). A proposito delle Ferrovie, lo voglio dire perché credo sia molto importante che l'Assemblea del Senato lo sappia, questa finanziaria dispone l'obbligo per le Ferrovie dello Stato di investire almeno la metà delle risorse alle stesse assegnate per infrastrutture locali e regionali e cioè a favore dei lavoratori pendolari e degli studenti. Credo stia sbagliando chi in questi giorni sta seminando sfiducia sui risultati che possono essere attesi da questa importante serie di misure, tutte mirate allo sviluppo della nostra economia, del nostro sistema industriale e produttivo, del nostro *welfare*. C'è un'altra parte della finanziaria di cui, per concludere, voglio parlare. Di quale sia l'efficacia reale delle misure dello sviluppo parleremo tra qualche mese, quando ne vedremo i risultati concreti e quando la maggioranza e il Governo potranno far valere fatti e numeri e potranno misurarsi con l'opposizione su basi chiare e non su *slogan* politici. Giorni fa, il Governo italiano, amici senatori, ha presentato a Bruxelles il Programma di stabilità ed ha preso l'impegno

Considero l'attenzione che il Governo Prodi ha riservato al debito pubblico, sia nella finanziaria che nel Programma di stabilità, il migliore segnale del cambiamento intervenuto nella politica economica del nostro Paese; lo considero il segno vero della svolta, la prova di voler seriamente sostituire al costume della cicala degli ultimi cinque anni una strategia seria che non pensi solo all'oggi, ma anche al futuro, al domani del nostro Paese. Voi sapete, signori senatori, che nel 2006 il debito pubblico ha pesato sui conti del nostro Paese per 72 miliardi di euro e che nel 2007 ci costerà ben 74 miliardi? Vi Vi ripeto: nel 2007 l'Italia pagherà 74 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Sapete che dal 1992 ad oggi gli interessi ci sono costati 1.200 miliardi di euro, senza che il debito scendesse neanche di un punto? Ecco, io mi chiedo e vi chiedo quale politica economica sia possibile per una Nazione i cui conti pubblici partono ogni anno con un *handicap* di un'entità molto più che superiore al doppio dell'intera manovra economica annuale. Un'ultima considerazione. Sappiamo che al 30 novembre scorso l'Agenzia delle entrate ha registrato maggiori versamenti rispetto all'anno scorso per ben 34 miliardi. Sappiamo che parte di queste maggiori entrate era già prevista ed impegnata, così come sappiamo che una parte dovrà necessariamente essere impiegata per onorare i nostri debiti. Sappiamo pure che è possibile che parte delle maggiori entrate non possa essere considerata strutturale e, conseguentemente, non possa essere utilizzata per grandi investimenti pluriennali. Detto questo e tutto ciò considerato, credo che sia possibile ad un senatore della maggioranza chiedere al suo Governo, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'economia, di valutare con attenzione se una parte anche limitata del maggior gettito - basterebbero 6-700 milioni non possa essere destinata a tre grandi obiettivi al cui raggiungimento è fortemente legato il valore politico di questa legislatura. Sto parlando della sicurezza pubblica, della ricerca scientifica e della scuola, degli aiuti ai cittadini non autosufficienti. Signor Presidente del Consiglio, se una parte delle nuove risorse andasse a questi tre obiettivi, la finanziaria per il 2007 ne risulterebbe straordinariamente rafforzata.

Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola in quest'Aula per invitare il Senato ad approvare la legge finanziaria e il bilancio che il Governo presenta e su cui chiede che gli sia rinnovata la fiducia. Da oltre ottanta giorni la manovra sui conti pubblici è oggetto di intenso lavoro nelle Camere elette dal popolo, viene discussa in ogni dettaglio sui giornali, alla televisione e nelle piazze. Il segno di quanto mi accingo a dire è espresso dalla stessa parola che dà il nome a questa procedura: fiducia. Fiducia nelle energie del Paese, nelle sue possibilità, nella capacità degli italiani di distinguere i fatti veri dalle false rappresentazioni, di udire le voci argomentanti anche attraverso il frastuono. Si usa dire che la politica è l'arte del possibile, ma è stato anche detto che la politica deve rendere possibile ciò che è necessario. Abbiamo cercato di farlo e abbiamo la profonda convinzione, conoscendo l'Italia e gli italiani (quelli che parlano e quelli che tacciono, quelli che lavorano e quelli che si preparano al lavoro) che, operando per il meglio nella difficile situazione ereditata, stiamo preparando per il Paese un futuro più sereno e costruttivo del presente e che questo sarà riconosciuto. Nessun atto di Governo, e tanto meno la legge finanziaria, che dell'attività del Governo costituisce un elemento fondamentale, può essere valutato senza rapportarlo da un lato ai fatti, dall'altro agli obbiettivi. Poiché è stato detto, ripetutamente, che questi fatti e questi obiettivi non sono stati comunicati in modo chiaro, cercherò di farlo di nuovo nel modo più sintetico in questa sede, che è la massima sede istituzionale e costituzionale per il Governo. I fatti che ci siamo trovati davanti sono semplici. L'Italia ha accumulato negli anni un debito pubblico esorbitante, immenso, con pochi paralleli al mondo: 1.600 miliardi di euro; per pagarne gli interessi, occorre reperire ogni anno 70 miliardi. Dal 2005 il peso di quel debito ha ricominciato a crescere più rapidamente della produzione nazionale, ciò che non era più avvenuto dal 1994. Senza l'euro e senza la ritrovata stabilità dei prezzi, due obbiettivi faticosamente e meritoriamente raggiunti dal I Governo Prodi, il peso degli interessi sarebbe insostenibile. I buoni del Tesoro vengono sottoscritti in larga parte dal mercato internazionale dei capitali. Se i conti dell'Italia fossero giudicati poco affidabili - e ancora oggi siamo sull'orlo di questo giudizio la legge del mercato imporrebbe un rialzo dei tassi, altrimenti i titoli dello Stato italiano resterebbero non collocati. Un solo punto in più di interessi sul debito aggrava la spesa pubblica di 15 miliardi di euro: un punto del prodotto interno lordo; ogni anno, non *una* *tantum*. Questo è il semplice fatto da cui partire; questo è il fatto troppo spesso taciuto nelle discussioni delle ultime settimane. Ecco perché l'azzeramento dell'avanzo primario, perpetrato nella legislatura passata dal precedente Governo, è un fatto di straordinaria gravità. Si è distrutto in pochi anni quanto si era faticosamente costruito in molti anni. In un Paese meno indebitato il fatto non sarebbe troppo grave; lo è in Italia per le ragioni dette. In passato, prima dell'euro, la soluzione era semplice: si creava inflazione e si svalutava. Quella che Luigi Einaudi chiamava la tassa più ingiusta era il rimedio perverso per tirare avanti. Oggi, fortunatamente, questo rimedio non è più possibile. L'avanzo primario è il saldo dei nostri conti al netto della spesa per interessi; è l'ossigeno, la riserva per poter onorare i debiti e pensare al futuro; è il risparmio della collettività. Come una famiglia, come un'impresa, anche la collettività deve amministrarsi guardando al futuro e non solo al presente. L'accumulo eccessivo dell'indebitamento è, prima di tutto, miopia, egoismo, sacrificio del benessere di domani al benessere di oggi, l'espropriazione dei figli e dei nipoti; è peggio della condotta della cicala, che nella favola non accumula debiti, ma si limita a consumare l'esistente. Come correre ai ripari? Nell'enunciazione la risposta è semplice: si rimedia mettendo a posti i conti, non perché ce lo impone l'Europa, ma perché ce lo impongono la salute pubblica, l'interesse nazionale e l'elementare buon senso. Questa risposta è stata annunciata nel giugno scorso dal Governo, che ha indicato anche le quantità necessarie allo scopo. Il disegno di legge finanziaria, che state per votare, raggiunge l'obiettivo di risanare i conti evitando il collasso finanziario del Paese al quale eravamo esposti? La risposta, di nuovo, è semplice: sì, l'obiettivo di risanare i conti viene raggiunto. Con una manovra per la massima parte strutturale viene, in un colpo solo, ricostituito un avanzo primario che già nel 2007 raggiungerà il 2 in un solo anno viene riportato sotto il 3 per cento il disavanzo che da quattro anni era superiore ai parametri europei e che, in assenza di interventi, si sarebbe collocato a valori prossimi al 4 Viene così rispettato l'impegno assunto dal precedente Governo al termine della passata legislatura. Anche su questo fatto si è troppo taciuto nelle ultime settimane. Non è stato facile mettere a punto le misure necessarie per il risanamento. Nonostante la presenza, nella maggioranza che ha vinto le elezioni, di culture politiche molto lontane tra loro nella loro genesi, l'obiettivo è stato raggiunto. La pluralità delle voci si è tradotta nell'omogeneità dei comportamenti. Che l'intero schieramento della maggioranza abbia condiviso le responsabilità e le scelte necessarie per governare in una situazione difficile qual è la nostra è un fatto d'importanza storica per l'Italia: un fatto che sembra passare inosservato. Se ci fossimo limitati, per la legge finanziaria del 2007, a fotografare il tendenziale, se non avessimo modificato nulla rispetto alle disposizioni della finanziaria precedente, sarebbero accadute quattro cose: in primo luogo, saremmo andati sotto di ben 15 miliardi di euro rispetto all'impegno assunto dal Paese nel 2005 per rientrare nei parametri di sana gestione sottoscritti nei Trattati. In secondo luogo, avremmo dovuto rinunciare a interventi di spesa essenziali, bloccando le ferrovie, interrompendo i lavori per le strade, sospendendo le missioni di pace; avremmo potuto rinnovare i contratti per l'impiego pubblico, e così via. luogo, avremmo dovuto rinunciare a ogni intervento di stimolazione dell'economia e dell'innovazione. In quarto luogo, avremmo dovuto rinunciare a forme di sostegno alle famiglie con figli, alle donne lavoratrici, agli anziani bisognosi ed altro ancora. Risanamento, sviluppo, equità. Per soddisfare queste quattro esigenze occorrevano risorse. Come reperirle? Le sole due vie possibili sono evidenti: ridurre le spese e aumentare le entrate. È vera l'affermazione, che si continua a ripetere quasi ossessivamente, che questa finanziaria opera solo sulle entrate e non fa nulla sulle spese? La risposta anche qui è chiara: l'affermazione è semplicemente falsa. Basta leggere le cifre per quello che sono. Questa finanziaria attua un contenimento della spesa corrente che ha pochi precedenti nel passato e rappresenta una vera e propria inversione di rotta rispetto alle tendenze in atto. Si ferma un treno in corsa e lo si fa operando sul motore, non solo sul freno. Lo si fa con misure permanenti, strutturali; non con palliativi da escogitare ogni anno di bel nuovo. Per la prima volta, si mette un vincolo all'aumento, sinora quasi incontrollato, della spesa sanitaria e questo - si noti - in accordo con le Regioni. Per la prima volta, si imbocca, concordandolo con essi, un *iter* di razionalizzazione della spesa dei Comuni. Le due misure introducono elementi importantissimi di federalismo fiscale, da tempo auspicati, ma non attuati sino ad oggi: al federalismo proclamato per una legislatura subentra il federalismo praticato. Sulle spese dei Ministeri si effettuano, più che in ognuna delle precedenti manovre di bilancio, risparmi sostanziali, eliminando - ove possibile - il superfluo. E altro ancora. Il tutto per un somma complessiva di oltre 10 miliardi euro. Un intervento pur tanto rigoroso non poteva, tuttavia, bastare, né per l'economia, né per la crescita, né per l'equità. Per l'economia occorreva rifinanziare ferrovie e opere pubbliche che, tra l'altro, rappresentano sostegni all'occupazione: circa 4 miliardi. Per l'economia e per la crescita occorreva alleggerire il costo del lavoro, così da rendere più competitive le nostre imprese: il cuneo fiscale costerà nel 2007 circa 5 miliardi, una parte dei quali andrà in busta paga. Per l'equità occorreva sostenere le famiglie e il lavoro femminile, i disabili e gli anziani indigenti; occorreva far pagare qualcosa di meno a chi guadagna di meno. Dunque, maggiori spese pubbliche, certo, ma anche spese pubbliche necessarie, spese d'investimento e spese per infrastrutture. Spese necessarie a conseguire obiettivi essenziali di efficienza e di crescita. La ricerca e l'università, certo meritevoli in futuro di investimenti ulteriori, sono comunque i comparti nei quali si è fatto ogni sforzo possibile per non pregiudicare gli investimenti. Rispetto all'evoluzione che si sarebbe avuta in assenza di interventi, si attua una ricomposizione e riqualificazione importante della spesa corrente, che viene ridotta, e di quella in conto capitale, che viene sostanzialmente incrementata. Anche questo fatto è stato quasi del tutto ignorato nella discussione delle ultime settimane. Vengo alle entrate. Sul fronte delle entrate si è puntato anzitutto al recupero dell'evasione fiscale: far pagare le tasse a chi non le paga. Nel valutare la pressione fiscale, l'aumento delle entrate derivanti dal ridursi dell'evasione è cosa ben diversa dall'aumento delle aliquote legali di prelievo. Non dispiaccia, questa affermazione, a chi non ama sentirla ripetere: la ripeto per rispetto ai tantissimi italiani che fanno il loro dovere di contribuenti onesti. La lotta all'evasione significa, in primo luogo, distribuire più equamente il carico tributario, non significa aumentarlo. Ed è stato proprio il Senato a tradurre in norma l'impegno politico più volte enunciato dal Governo di ridurre le aliquote di prelievo allorché la lotta all'evasione abbia prodotto un permanente aumento delle entrate. L'evasione, che in Italia è patologia allo stato epidemico, può venir progressivamente arginata e ridotta a patologia sporadica. Non certo con i condoni. Al contrario: con politiche fiscali tenaci e continue, come quelle che abbiamo intrapreso. I primi risultati già si vedono, altri verranno. Quando saranno consolidati, si spera in tempi brevi, si potrà finalmente cominciare a far diminuire le aliquote. Un'altra parte delle risorse necessarie per la crescita viene dall'impiego di una parte (la sola parte che i lavoratori liberalmente decideranno di non assegnare alla previdenza integrativa) del trattamento di fine rapporto delle imprese con più di 50 dipendenti. Questa misura non toglie assolutamente nulla né alle imprese, né ai lavoratori, come ha spiegato lucidamente una voce isolata su un quotidiano di cui è editore proprio la Confederazione degli industriali. I soldi sono e restano dei lavoratori e l'INPS si limita ad investirli in infrastrutture per raggiungere scopi largamente condivisi. Dove sta lo scandalo? Un fuoco di paglia violento e fatuo. La riprova è che del TFR da qualche settimana non si parla più. Invece, la pressione tributaria (le tasse sui cittadini e le imprese che già adempiono al loro dovere fiscale) viene ridotta già in questa finanziaria, se si tiene conto del complesso delle misure adottate. Aumentano sì i contributi previdenziali, ma (particolarmente col passaggio al sistema contributivo che è in corso) i contributi previdenziali rappresentano un risparmio dei lavoratori che verrà loro restituito in forma di maggiori pensioni future e non sono quindi assimilabili alle tasse in senso stretto. L'aumento è necessario, non solo per assicurare l'equilibrio del sistema nel lungo periodo, ma anche per migliorare le pensioni future dei giovani. Nel complesso, l'aumento del prelievo aggiuntivo sul settore privato rappresenta una quota modestissima della manovra complessiva. È, questo, un altro dato di fatto troppo spesso trascurato dall'analisi cui la manovra finanziaria è stata sottoposta in queste settimane. Si sarebbe potuto procedere ritoccando un solo comparto, ad esempio alzando l'IVA; la Germania della grande coalizione l'ha alzata di tre punti. Questa scelta è stata scartata per non creare intralci ai consumi e alla crescita. Si è preferito rimodulare, con mano leggera, una serie di comparti allo scopo di coniugare la cura per la crescita con quella per l'equità. Chi ha parlato ossessivamente di un rialzo generalizzato dell'imposizione fiscale, di 67 nuove tasse, ha deliberatamente ignorato questi dati, i quali non si annullano certo per il fatto di venir contraddetti a parole una, cento o mille volte nei messaggi televisivi. La procedura che in Italia conduce all'approvazione della legge finanziaria è ben nota e praticata da anni. Questa volta, però, essa ha attraversato in sei mesi vicende a dir poco inconsuete, per non dire eccezionali, sulle quali non si può sorvolare. Nessuna finanziaria precedente ha conosciuto un *iter* così trasparente e così intensamente partecipativo quanto l'attuale. Ogni Ministro ha preso parte al gigantesco cantiere, manifestando esigenze raccolte nel concreto contatto con la realtà della quale è il responsabile politico e istituzionale di punta. Le Regioni, le Province, i Comuni, le rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori, i commercianti, gli artigiani sono stati ascoltati a lungo, ripetutamente, approfonditamente. Il Governo ha operato una sintesi e l'ha espressa in tre punti: sviluppo, risanamento, equità. Le molte centinaia di disposizioni che compongono la manovra sono state più volte sezionate, riconsiderate sulla base di critiche e osservazioni, rimodulate, riscritte. Il Parlamento, a sua volta, ha introdotto modifiche, miglioramenti, elementi ulteriori, pur lasciando intatte le mura portanti della manovra. Tutto questo è positivo, è espressione di democrazia, è strumento per migliorare i testi legislativi, è acquisizione di apporti critici e di consensi. Guai a lamentarsene come se fosse un male del quale dovremmo liberarci. Lo dice un Ministro che non proviene dalla professione politica, ma che della politica, alla quale è stato chiamato, ha un altissimo concetto. È positivo, ma ha i suoi costi: il flusso ininterrotto delle notizie ha dato l'impressione - un'impressione spesso lontana dalla realtà - di affanno, di confusione, di incertezza. Me ne dolgo e me ne scuso, a nome del Governo, con i cittadini. A questo occorrerà porre rimedio, anche migliorando le procedure, per far sì che già dall'anno prossimo il percorso divenga più lineare. È naturale la tentazione di pensare a quanto sia più agevole e più gradevole la procedura dei Paesi nei quali la proposta del Governo va tal quale al voto del Parlamento. Il *budget* inglese viene approvato in cinque giorni e tuttavia anche in quel sistema l'intervento dell'Aula di Westminster avviene dopo un'intensa fase di lavoro e confronto parlamentare nella competente Commissione. Al riguardo, convengo pienamente sulle considerazioni svolte in questa sede dal presidente Morando, cui desidero rivolgere - così come al relatore alla Commissione, senatore Morgando - un ringraziamento particolare per l'equilibrio, la fermezza, la chiarezza di metodo con cui ha diretto i lavori. Chi vi parla è un fermo sostenitore della concertazione, del confronto, della ricerca della soluzione più accettabile in termini di equità e di efficacia ed è ben consapevole di quanto sia essenziale, sostanziale il contributo che deriva da un pieno coinvolgimento del Parlamento. Non tutto è però sempre positivo nel processo vitale e tormentato della nostra democrazia. E proprio per salvaguardare l'inestimabile valore di questo processo, occorre a tutti i costi evitare che la spinta, pur legittima, per la tutela degli interessi particolari superi la soglia del ragionevole. Occorre evitare che il coro delle richieste particolari, pur comprensibili e quasi sempre di per sé giustificate, diventi così assordante da far tacere la voce profonda ma fievole dell'interesse generale e del bene comune. Il rischio per l'Italia sarebbe molto alto, se si smarrisse la bussola dell'interesse generale. Lo ha detto benissimo Gustavo Zagrebelsky, in un articolo di pochi giorni fa, che cito «La politica pesca dalla società le istanze che essa vuole rappresentare. Tante cose eterogenee e tanti soggetti sociali, conflittuali tra loro e al loro stesso interno, che con i mezzi più diversi cercano di farsi strada e che la classe politica è tenuta a selezionare. Un caos di istanze tra le quali si deve però fare una prima, fondamentale distinzione, a seconda della prospettiva in cui si collocano: individuale e immediata, oppure generale e duratura. In questa distinzione traspare il pericolo della catastrofe della democrazia, cui è esposta per cecità o per incapacità di allungare il suo sguardo». il suo sguardo». Ebbene, è per l'interesse generale dell'Italia che si è fatta questa finanziaria. Il Governo ha ascoltato e raccolto diverse istanze, ma senza perdere di vista i tre obiettivi che ho appena ricordato e senza mancare il traguardo stabilito. Un traguardo, sia detto per inciso, che oggi alcuni contestano avanzando la tesi che l'intero aumento del gettito del 2006 sia ormai strutturale e, soprattutto, aggiuntivo rispetto alle previsioni. Non è vero. Il Governo ha costantemente aggiornato le stime del gettito e la finanziaria tiene conto, quasi per intero, del maggior gettito tributario del 2006. Non c'è quindi un tesoro nascosto da spendere, almeno per ora. Vi è chi ha sostenuto persino la tesi stravagante che per sistemare tutto sarebbe bastata una manovra da 15 o addirittura da 7 miliardi, una tesi del tutto fuori della realtà. Giudizi fondati su una lettura errata, se non pretestuosa, dei fatti e dei dati. Non l'albero, ma addirittura il cespuglio o il filo d'erba, ha nascosto la foresta. E allora non meravigliamoci se il cittadino non capisce. E magari protesta. Ma la foresta c'era, c'è, e a questa bisognava e bisogna guardare. In questi mesi di intenso lavoro è stata mia costante cura verificare, quanto più spesso possibile, le richieste e le reazioni di chi lavora e produce. Piuttosto e prima per ascoltare che per persuadere. Ciò mi è sembrato e mi sembra tanto più necessario in presenza di misure senza dubbio severe. Ebbene, in Veneto come in Lombardia, in Romagna, in Abruzzo, in Toscana e altrove ho ascoltato certamente critiche, insofferenze, impazienze. Ma anche, in misura non inferiore, segnali inequivocabili di consapevolezza e disponibilità a modificare comportamenti che pregiudicano uno sviluppo sano dell'economia, a cominciare dall'evasione fiscale. Quando confronto l'immagine catastrofista di tanti commenti con quella degli incontri pubblici e privati, allargati o ristretti, ai quali ho preso parte personalmente, non posso non notare uno iato, quasi si trattasse di due mondi separati. La mia convinzione, che ogni incontro sembra confermare, è che l'Italia ha in sé energie vitali ancora enormi. Certo, non vi è più la spinta prepotente al benessere che fu propulsiva negli anni Cinquanta e Sessanta, né la sfida immediata del Mercato comune che costrinse a fare subito il salto necessario a vincere la concorrenza dei Paesi vicini. Certo, oggi la sfida è più ardua e non può essere agevolata dallo strumento facile e ingiusto delle svalutazioni competitive. La sfida può e deve venire da una giusta ambizione sul futuro del Paese. Mi sia lecito rivelare, al termine di un processo politico intensissimo, durato sette mesi, che in più momenti ho temuto che si avverasse la sorte del vecchio pescatore raffigurato da Hemingway ed evocato da Altiero Spinelli nel febbraio 1984 davanti al Parlamento europeo: il rischio di giungere a riva con la sola lisca nuda e spoglia del pesce tanto faticosamente arpionato. La sorte, ma anche il merito dei tanti soggetti, politici e non, che hanno contribuito a costruire la finanziaria che ora siete chiamati a votare, hanno determinato un esito diverso. Ci sono, nella finanziaria e nell'azione complessiva del Governo in questi mesi, le premesse per costruire il domani. Innanzitutto una finanza pubblica più sana, condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile, per rinforzare la voglia di investire sul futuro, per orientare risorse pubbliche alla crescita e, soprattutto, per ridare prospettive ai giovani. Bisogna, quindi, essere fieri di quanto fatto fin qui e del coraggio del Governo nel dire la verità ai nostri concittadini, ma bisogna nello stesso tempo riconoscere che siamo solo all'inizio, che molto rimane da fare in tutti i campi che ho appena ricordato e che il lavoro andrà continuato, fin da subito, con ancor più tenacia e volontà. Questa finanziaria ci permette di farlo con rinnovato ottimismo. Vi ringrazio.

appena concluse tali dichiarazioni di voto e immediatamente prima del voto, il sottosegretario D'Andrea darà conto di questi aspetti che, ripeto, c'è stata premura di esaminare assieme ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione bilancio.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula (di quest'Aula e anche dell'altra Aula del Parlamento), preliminarmente, alcune considerazioni metodologiche. Siamo convinti che le modalità con cui approviamo la finanziaria, disciplinate da una legge del 1978, siano ancora oggi quelle che giovano all'azienda Italia, al nostro Paese, a questa maggioranza e a questa minoranza? operiamo, dal DPEF, emanato a giugno, fino alla finanziaria, approvata a fine dicembre, per dirla come ha detto un commentatore su un importante quotidiano stamattina, con la fiera degli emendamenti. In sei mesi, la nostra finanziaria vive sui giornali, vive con gli emendamenti che esistono e non esistono, che sono presentati e che sono ritirati; praticamente, per cinque o sei mesi bloccando di fatto l'attività del Parlamento. Ho colto, nell'intervento del ministro Padoa-Schioppa, un riferimento al *budget* inglese. Io credo che noi dovremmo avviare, qui, in modo *bipartisan*, da subito, una riflessione: ci conviene continuare con questo impianto, che è figlio di una legge del 1978, nella quale l'obiettivo da raggiungere era quello di fare in modo che le Commissioni bilancio di Camera e Senato governassero, probabilmente, più dell'Esecutivo, o è meglio orientarci in direzione del sistema di approvazione inglese, il *budget* cui faceva riferimento il ministro Padoa-Schioppa, o del sistema francese, che ritiene inemendabile la finanziaria e quindi, sottoposta al Parlamento, o passa o non passa? questo interrogativo al Parlamento perché credo che, se riuscissimo a superare l'attuale sistema di finanziaria, probabilmente i 1.365 commi, di cui abbiamo ascoltato in Aula e di cui abbiamo letto sui giornali, non capiterebbero più: 1.365 commi sono difficili per tutti a leggersi in due giorni; probabilmente dobbiamo aggiornarci. Per quanto riguarda invece il merito non ho difficoltà a dire che in Senato abbiamo migliorato il testo che ci era arrivato dalla Camera; mi confortano e supportano, tra l'altro, i dati riferiti dal ministro Padoa-Schioppa nel suo intervento: 1.600 miliardi di euro il debito pubblico dell'Italia; dato clamoroso: 70 miliardi di euro l'anno per pagare soltanto gli interessi sul nostro debito pubblico. Nonostante questa situazione così drammatica, nonostante questa situazione particolare dei conti pubblici, che come Unione abbiamo ereditato, siamo riusciti a fare una finanziaria di rigore, di equità e di sviluppo. Lo dico al senatore Azzollini, che faceva riferimento ad una finanziaria di rigore. Siamo riusciti a coniugare,

che gli italiani questo lo capiranno. Noi dell'Italia dei Valori apprezziamo particolarmente, in questa finanziaria, la connotazione che essa ha con riferimento all'evasione fiscale, la connotazione che essa ha sul contenimento dei costi della politica, la connotazione che essa ha circa forme più avanzate di liberalizzazione e la connotazione che ha su forme ancora più avanzate di solidarietà. Ma, allo stesso tempo, affermiamo che si poteva fare qualcosa in più. Notiamo ancora timidezza sulle liberalizzazioni e - consentitecelo, signor Ministro e amici della maggioranza - notiamo ancora timidezza sui costi della politica. Noi voteremo questa finanziaria; la voteremo intendendola, però, come un punto di partenza. *(Richiami del Presidente)*. È la prima di cinque finanziarie; crediamo che gli italiani capiranno, però occorre che la ripartenza, da subito, sia visibile e percepibile.

un nuovo approccio alle politiche economiche e sociali dell'Italia ed un nuovo modo di gestire la finanza pubblica e di concepire un utilizzo più strategico delle pubbliche risorse. Dopo l'esperienza appena conclusa del Governo di centro-destra, l'Italia è chiamata ad imboccare la via del recupero in un contesto comunitario ed internazionale corroso, purtroppo, dalla logica di un mercato senza regole e che ha ripiegato su se stesse le potenzialità nazionali dei Paesi a forte tradizione occidentale, chiamate a misurarsi con la globalizzazione sempre più evidente e marcata. Paese può svolgere, se lo vuole, un ruolo di primissimo piano per le potenzialità che esprime, per la ricchezza, che è sotto gli occhi di tutti, in termini di nuova impresa e di nuova capacità di comprendere a pieno il vento comunitario e globale che ci sta davanti e che esige, da parte dei governanti, linee certe e comportamenti di governo rigorosi. In questo contesto la manovra definita dal Governo Prodi, con la regia del ministro dell'economia Padoa-Schioppa, rappresenta un misto di rigore e di prospettiva per la nostra economia e, soprattutto, rappresenta un punto di partenza rispetto alle sfide della liberalizzazione liberalizzazione e di un mercato sempre più esigente, che pone a ciascuno di noi il dovere di coniugare la risposta allo Stato sociale anche con la tenuta dell'area di imprenditoria liberale, corrosa da un appesantimento fiscale senza ragione e senza limiti. In tal senso, va interpretata una nuova filosofia delle politiche economiche, che vanno proiettate in direzione di un recupero della centralità dello Stato sociale, senza perdere di vista la funzione salvifica che l'imprenditoria

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tre brevi punti. Primo: in sede di Commissione finanze e tesoro, il 28 novembre scorso, ho rappresentato l'esigenza di una sostanziale revisione della procedura di bilancio, alla luce delle esperienze dell'ultimo decennio. Ho anche auspicato più penetranti verifiche dei risultati dei principali provvedimenti assunti. Per questo sono favorevole a che abbiano seguito le specifiche proposte avanzate in quest'Aula dai senatori Morando e Azzollini. Secondo punto: oggi l'economia italiana sta attraversando un momento delicato e importante. Per troppi anni, la crescita economica è stata sensibilmente inferiore sia al nostro potenziale di sviluppo sia alla media dell'Unione Europea e questo in presenza di una forte espansione dell'economia mondiale. Da qualche mese, la nostra economia sta manifestando segni di risveglio. È di interesse generale trasformarli in crescita robusta, far sì che l'apparato produttivo riconquisti un ritmo costante di incremento della produttività e divenga così più competitivo sui mercati interni e internazionali. Solo con la crescita, con lo sviluppo, le giuste aspirazioni degli italiani potranno trovare soddisfacimento. So bene che, per conseguire una crescita robusta, cioè elevata e duratura, è necessario riequilibrare i conti pubblici. So bene, altresì, che non è facile nella manovra di bilancio conciliare due obiettivi: crescita e stabilità. La presente legge finanziaria si propone di conseguire ambedue questi fini. Quel che so per certo è che sarebbe dannoso per l'economia italiana e provocherebbe conseguenze negative sui mercati entrare nel nuovo anno in regime di esercizio provvisorio per la mancanza dei documenti finanziari fondamentali per il funzionamento dello Stato. È dal 1988 che si è evitato il ricorso all'esercizio provvisorio. Darò quindi il mio voto favorevole alla legge in esame. Non posso, infine - ed è il terzo punto - non rimarcare, con disappunto, che ancora una volta viene fatto ricorso ad un modo di legiferare che, non da oggi, ritengo improprio. Articoli di legge composti da una innumerevole quantità di commi, in questo caso oltre mille, è un modo di procedere che occorre dismettere. *(Applausi

più giovani, si ricordano i film dell'epopea di Little Big Horn e di «Ombre rosse». Non considero certamente né l'amico Matteoli né l'amico Schifani, capi di tribù indiane, ma stasera, prendendo la parola per dichiarare che voterò a favore, parlo con lo spirito temerario di un giovane ufficiale del 7° Cavalleria che va alla carica temendo di finire a Little Big Horn, ma sperando di soccorrere John Wayne in «Ombre rosse». Dichiaro che voterò, non senza riserve e preoccupazioni, a favore della legge finanziaria su cui il Governo ha posto legittimamente la fiducia. Voto a favore, con serie riserve dal punto di vista giuridico e della correttezza politica, poiché formulare un maxiemendamento di 1.365 commi - non me ne abbia il Ministro dell'economia - è insieme ridicolo e aberrante. Se il voto di fiducia fosse un contratto tra i senatori rappresentanti del popolo e il Governo, esso sarebbe certamente invalido: invalidato dall'ignoranza (perché mi chiedo quanti senatori sappiano su che cosa votano; io non lo so) e dalla mancata approvazione espressa delle clausole vessatorie. Voto a favore, con preoccupazione, perché la legge finanziaria dimostra quanto forte sia la conflittualità interna al Governo e alla maggioranza, per superare la quale, con mia grande meraviglia, nella fase finale, come mi ha detto più di un Ministro, il maxiemendamento non è stato né sottoposto al Consiglio dei ministri né fatto conoscere preventivamente ai membri del Gabinetto. Forse siamo transitati verso il Governo del *Premier* e non più verso il Governo collegiale, come previsto dalla Costituzione. E dimostra anche la mancanza di una vera e seria linea di politica economica e sociale, che, dopo le proteste di tutte le categorie, solo la presenza nella maggioranza e nel Governo della benemerita - per questo Governo - sinistra radicale, cui fanno riferimento i movimenti, e l'acquiescenza politica dei sindacati confederali, salva dalle manifestazioni di piazza anche, magari, con «violenza a bassa intensità». Nonostante tutto questo, voterò a favore della fiducia e quindi per l'approvazione della legge finanziaria, e poi anche della legge di bilancio, anche se essa ha ormai perduto i suoi propri caratteri costituzionali di legge formale e di semplice autorizzazione all'erogazione della spesa e alla riscossione delle entrate. Voto a favore perché la mancata approvazione di queste due leggi getterebbe il Paese nel caos e sfregerebbe il volto già ferito dell'Italia in Europa e nella comunità internazionale.

si rifiutò di far ricontare le schede, perché, si disse, il popolo e l'opinione pubblica avevano accettato la votazione. Come è accaduto in America: Kennedy era stato sconfitto e fu accettato; certamente Bush probabilmente era stato sconfitto e l'avversario riconobbe l'esito. E poi, cosa vogliamo: il mite, mio amico, Ministro della difesa

con lo spirito del temerario ufficiale subalterno del generale Custer, sperando che il Paese vada, non a Little Big Horn ma alla liberazione della diligenza con John Wayne, dichiaro di votare a favore

la mia posizione personale, come quella dello schieramento di cui faccio parte, non può che essere fortemente critica, non solo innanzi al nuovo testo presentato, ma per l'intero comportamento tenuto da questo Governo in questi giorni così particolari. Non mi soffermerò a spendere ulteriori parole, oltre quelle già pronunciate da altri miei colleghi, sulla irritualità nella presentazione del maxiemendamento, sulla violazione di numerose norme sia costituzionali che del Regolamento del Senato e sulla ennesima richiesta di fiducia di questa traballante maggioranza in pochissimi mesi dal suo insediamento. Un modo di agire, questo, totalmente sconsiderato e deleterio per l'intero Paese. Oggi, infatti, ci viene qui richiesto (e mi rivolgo tanto alla maggioranza quanto all'opposizione) di esprimere un voto, espressione della volontà popolare di cui siamo portatori, senza aver avuto - ha ragione presidente Cossiga - un testo così complesso in tempo per rendergli veramente giustizia. Sin dalla sua originaria presentazione, questa finanziaria, la prima del Governo Prodi, ha mirato a operare una manovra di ben 35 miliardi di euro, andando a incidere sulle famiglie italiane per 5,5 miliardi di euro, pari a una media di 251 euro per nucleo familiare. Con la proposizione di questo nuovo testo noi tutti speravamo in una presa di coscienza da parte della maggioranza, anche alla luce degli enormi dissensi raccolti durante la manifestazione del 2 dicembre, ma abbiamo ancora una volta constatato il sostanziale fallimento degli obiettivi annunciati e mai perseguiti nella realtà. Un altro treno e stato perso. Con questo nuovo provvedimento non è stata modificata l'ossatura della manovra, che è e rimane una manovra di tasse, una manovra oppressiva, che chiede ai cittadini ulteriori sacrifici senza offrire altrettanti servizi. C'è da domandarsi se realmente questo Governo si aspetti la gratitudine dai cittadini o di intere categorie. Di certo non ringrazieranno tutti coloro che posseggono un'abitazione (l'82 per cento degli italiani) e che speravano nell'eliminazione dell'odiata ICI, e invece la vedranno aumentare insieme agli estimi catastali. Non ringrazieranno gli operatori delle scuole parificate, frequentate dai nostri figli, che si vedranno erogare somme relativamente inferiori rispetto a quelle destinate, ad esempio, al «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati» per la scolarizzazione dei propri figli. Non ringrazieranno il milione circa di motociclisti verso i quali è stata usata la mano pesante, soprattutto per quelli intuitivamente meno abbienti, che non hanno la moto nuova, e per i quali la tassa di possesso è aumentata addirittura del 100 per cento. Non ringrazieranno i milioni di famiglie che si trovano a dover sostenere i canoni di locazione del proprio immobile, quasi ignorati da questo provvedimento nonostante le nostre proposte che miravano alla possibilità per le famiglie di detrarre parte dell'onere per la casa o all'introduzione di un'aliquota unica, che prevedeva per i redditi derivanti dalla locazione di immobili un'imposta sostitutiva di quelle sui redditi con aliquota unica del 20 per cento. Come non ringraziano gli atenei italiani, che da tempo denunciano la chiusura del Governo a ogni dialogo. Non ringrazieranno gli avvocati, i notai, i commercialisti, come tutti i professionisti; non ringrazieranno gli operai, gli operatori turistico-portuali, che in questi giorni hanno tentato di far sentire la propria voce. E si prepara a non ringraziare, egregio Presidente, tutto l'associazionismo cattolico. Non ringraziano, come ho detto, larghe fasce della stessa maggioranza (un plauso va al collega Salvi per il discorso fatto questa mattina, politicamente e intellettualmente onesto). Ma allora, mi domando, chi voterà questa finanziaria? A questo proposito, cito una preoccupazione che viene ancora da un altro settore, dal mondo dei rettori delle università, e, nella fattispecie, da Azione universitaria, che, in una lettera indirizzata alla senatrice Levi-Montalcini, dice testualmente: «Sappiamo che al Senato il voto della senatrice a vita potrebbe essere determinante, ma siamo anche convinti che il suo amore per la scienza e per l'università sarà superiore alle pressioni politiche che riceverà in queste ore». Non commento. In questa finanziaria non si è voluto incidere sulle spese pubbliche per non privare il proprio serbatoio di privilegiati delle risorse promesse sotto campagna elettorale. Si è cosi pensato di aumentare la pressione sui cittadini. Ringrazieranno invece le grandi banche e il loro sistema, per i grandi guadagni che avranno per via della necessità di tutti i cittadini, che non vogliono essere perseguitati dal fisco, di aprire i conti in banca, anche le nostre nonnine, le nostre zie, gli anziani che non sanno cosa sia una carta di credito. «C'è un pasticcio e una confusione che a noi non piacciono. Stiamo andando verso la fine di questa situazione ormai insopportabile di un documento finanziario che dura da tanto tempo. Credo che il bilancio, al di là delle luci e delle ombre, bisogna verificarlo in modo che il prossimo anno non sia così». Non pensiate che questa sia una mia affermazione dal pulpito dell'opposizione: l'ha detto oggi a Napoli Raffaele Bonanni, segretario della CISL. D'altronde, ne ha ben donde ed è libero di farlo, come del resto liberi di farlo sono tutti i sindacati in sciopero pressoché costante durante il Governo Berlusconi, accusato di non concertare ma di consultare. Il passo in avanti, al contrario delle promesse elettorali, che oggi fa il Governo Prodi è quello che non concerta e non consulta; e anche qui qualcuno potrebbe dire che questi sono soltanto esercizi dialettici di opposizione. E allora cito Prodi, che ieri su «la Repubblica» «La mia colpa e di non aver tra l'altro, consultato nessuno, né imprese, né sindacati, né artigiani». E io aggiungo, Presidente, purtroppo neanche i cittadini italiani nella loro interezza. Dov'è finita la tanto proclamata equità? Dove sono le riforme strutturali tanto sbandierate? Dove gli incisivi interventi in tema di occupazione? Forse si è inteso giocare sulla frettolosa presentazione di questo provvedimento, in modo che ne fosse celato il vero intento, cioè quello di reinstaurare una centralità dello Stato controllore e oppressore, nemico, da eludere, da aggirare. Un nemico che viola le sue stesse leggi, basti pensare alla più volte elusa norma che proibisce la retroattività delle disposizioni tributarie. Non voglio dare *ultimatum*, perché non posso, ma Antonio Di Pietro sì, lui è Ministro di questo Governo ed è un costruttore di questa finanziaria che dice testualmente: «Io sto con gli italiani» - anche noi, Ministro - «che sono stufi di sentire di formule e formulette, centri e centrini, destra e sinistra, fase 1, 2 e 102. Le azioni furbesche di qualcuno all'interno della maggioranza e forse anche del Governo, che ha inserito negli emendamenti un provvedimento disastroso per la credibilità dell'Unione, che è quello della prescrizione di fatto per i reati contabili commessi dalla Corte dei conti. È un emendamento che porta l'Unione a comportarsi alla Berlusconi». Magari, signor Ministro: se così fosse, tutte le categorie da me citate all'inizio del mio discorso avrebbero sì ringraziato il Presidente del Consiglio. Vado alla conclusione, signor Presidente. Avendo citato tutto l'arco della maggioranza, non prima del grido di dolore dei cittadini italiani, non poteva infine mancare il più autorevole ministro di questo Governo, Giuliano Amato, che dice: «Posso collocarmi anch'io tra gli scontenti della legge finanziaria» - mi spiace, Ministro, non c'è più spazio, siamo in troppi - «Mi auguro che il Senato la cambi. Se non succede, da Ministro avrei ragioni per protestare». Ministro, ci abbiamo provato noi a cambiarla, ma la sua maggioranza non ce l'ha consentito. Sia conseguente a ciò che ha affermato e voti no insieme a noi. Con noi c'è tutto il Paese, Ministro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo consapevoli che questa legge finanziaria, forse come mai finora, ha avuto puntati addosso i riflettori del Paese, facendo discutere, polemizzare e scendere in piazza milioni di cittadine e cittadini e non solo di destra. Non c'è dubbio: sulla finanziaria abbiamo un problema di consenso. Dobbiamo prendere atto del malcontento di queste ultime settimane, rifletterci e sforzarci di capirne le ragioni. Ciò non toglie che restiamo fermamente convinti della bontà degli obiettivi di questa manovra; ed insieme al presidente del Consiglio Romano Prodi e al ministro dell'economia Padoa-Schioppa siamo anche noi certi che i cittadini cambieranno opinione non appena il Paese comincerà nuovamente a crescere. Ho già detto in sede di votazione del decreto fiscale - e lo ripeto - che il Governo avrebbe dovuto illustrare ai cittadini, senza mezzi termini, l'eredità pesante lasciataci dal Governo di centro-destra. Sin dalla campagna elettorale avrebbe dovuto denunciare la catastrofica situazione economica del Paese: il debito pubblico

Questo debito pesa soprattutto sull'economia, sul mondo imprenditoriale, perché mancano le risorse in conto capitale per i grandi investimenti e per migliorare i fattori di produttività. L'Italia non può permettersi di essere e di rimanere il fanalino di coda dell'Europa. Anche la gestione di questa finanziaria e del bilancio è stata criticata dai cittadini e dai colleghi in quest'Aula, in quanto troppo confusa. Ma, a differenza del passato, questa finanziaria nel suo *iter* parlamentare - ed è bene che così sia stato rivalutato il Parlamento - ha avuto come linea guida la ricerca di consenso e di concertazione, prima con le parti sociali, poi con il Parlamento stesso. La bozza iniziale, in parte criticata giustamente, in parte criticata per motivi strumentali, ha mantenuto fermi i suoi obbiettivi, ma - va detto a chiare lettere - è stata profondamente migliorata, specialmente in Commissione bilancio. Cari colleghi, dobbiamo riconoscere lo straordinario lavoro di confronto tra maggioranza e Governo nella «cabina di regia» e poi nella Commissione competente anche tra maggioranza ed opposizione. Ringraziamo il presidente Morando e il relatore Morgando per il grandissimo sforzo che hanno compiuto. Questo lavoro, parso ahimè confuso agli occhi dei cittadini, alla fine ha contribuito, ripeto, specialmente qui in Senato, a migliorare il testo senza stravolgere gli obiettivi di equità sociale e di crescita. Questa, infatti, è una finanziaria che vuole far ripartire il motore della ripresa e del rilancio dell'economia. Una finanziaria che punta a liberare risorse per favorire la crescita, superando anni di stallo. Una finanziaria che promuove lo sviluppo per riconquistare la fiducia degli altri Paesi europei e dei mercati internazionali; e ci sta pian piano riuscendo: la manovra ha già ottenuto l'approvazione dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea e persino dal severissimo Fondo monetario internazionale. Questa manovra riuscirà a riportare il *deficit* sotto il 3 per cento del PIL, rispettando pertanto gli impegni presi con l'Unione Europea. È partita finalmente una strategia di bilancio in favore della crescita, dopo anni di perdita di competitività e politiche che non sono riuscite a spingere lo sviluppo. Questa è una finanziaria con cui l'Italia incomincia a risanare i conti pubblici e a lavorare sulla crescita; ripeto: sulla crescita. L'opposizione

Ma non ci si può fermare solo al pagamento dei debiti: servono anche risorse per la ricerca, l'equità sociale e lo sviluppo economico. Questo fa la finanziaria con l'altra metà A dispetto di chi punta l'indice su una regia della sinistra massimalista e dei sindacati, questa finanziaria punta sulla produttività, che mai è stata così centrale negli obiettivi dei Governi degli ultimi decenni. È infatti una manovra che, con i miglioramenti apportati alla Camera e al Senato, ha introdotto importanti misure a favore delle piccole e medie imprese. Ricordo la riduzione dell'IRAP, che abbasserà i costi del lavoro. Ricordo i trasferimenti di azienda, che fino al terzo grado saranno esenti da tasse di successione e donazione; anche il nostro Gruppo si è impegnato fortemente su questo, ed è un grande

dei contributi previdenziali per gli apprendisti artigiani è stata ridotta per i primi due anni. Ricordo, infine, gli studi di settore e le società di comodo resi meno pesanti. E tutto ciò non a scapito delle famiglie e del settore sociale. Si pensi al forte impegno del Governo a rimodulare la curva IRPEF a favore delle famiglie, soprattutto di quelle numerose; all'estensione degli assegni familiari ai nuclei numerosi; alle franchigie per successioni e donazioni per coniugi ed eredi in linea diretta, fratelli e sorelle e soggetti portatori di *handicap*. Ricordo, poi, l'importantissimo impegno del Governo, preso qui al Senato, ripreso nell'articolo 1 di questa finanziaria, condiviso da tutta l'opposizione, ossia di usare le maggiori entrate, derivanti dalla lotta all'evasione fiscale dopo gli obiettivi di risanamento - alla riduzione della pressione fiscale a favore di chi paga le tasse, dando priorità a misure di sostegno del reddito dei soggetti incapienti. Sempre al Senato, grazie alla nostra proposta come Gruppo Per le Autonomie, abbiamo dato un ulteriore *input* ad un tema importante, quale quello dell'avvio delle pensioni integrative.

l'avvio delle pensioni integrative e anche l'anticipazione della riforma del TFR al 2007 e, con l'inizio del prossimo anno, ritengo sia opportuno, nonché doveroso nei confronti delle nuove generazioni, dei giovani, che Parlamento e Governo mettano mano alla stagione delle riforme, partendo proprio da quella del sistema pensionistico. Credo che l'allungamento dell'età pensionabile non debba essere obbligatorio, ma possa benissimo essere promosso da un sistema di incentivi che premi chi vuole vuole rimanere al lavoro. Devono poi seguire ulteriori riforme strutturali che coinvolgano tutti i settori, iniziando dalla pubblica amministrazione. Invitiamo a spingere soprattutto sul fronte delle liberalizzazioni ed auspichiamo - lo sottolineo - lo sviluppo del federalismo fiscale per trasferire alle Regioni e alle Province la responsabilità non solo per le uscite, ma anche per le entrate. Le stesse verrebbero così responsabilizzate maggiormente. la bozza originale della manovra andava fortemente modificata e lo abbiamo fatto. Abbiamo apportato modifiche importanti per promuovere le piccole e medie imprese, le famiglie, la ricerca e la cultura. Siamo anche soddisfatti - e vorrei ringraziare il Governo - per l'accoglimento di un serie di modifiche migliorative promosse dal nostro Gruppo. Pertanto, annuncio che il Gruppo Per le Autonomie esprimerà la fiducia a questo provvedimento e a questo Governo.

intervengo per annunciare la fiducia e il voto favorevole del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani

Vorrei recuperare questo tempo, Presidente.

dopo il passaggio al Senato. È migliorato sul piano sociale e sul piano della redistribuzione. C'è un cambiamento di segno importante rispetto al passato: c'è più equità e più sviluppo. Il sistema delle imprese, attraverso la riduzione del cuneo fiscale, può essere reso più competitivo sui mercati internazionali; vi sono gli incentivi automatici per la nuova occupazione e per gli investimenti. Avevamo detto che era necessaria una finanziaria di risanamento, equità e sviluppo: di risanamento, perché abbiamo trovato una situazione dei conti pubblici pubblici più difficile rispetto alle previsioni. Ci siamo accorti in queste settimane, per esempio, del nuovo buco nel sistema di finanziamento dell'Alta Velocità ferroviaria.

Con la rimodulazione delle aliquote fiscali, i redditi fino a 40.000 euro beneficeranno di una riduzione del carico fiscale e, insieme alle nuove misure sulle detrazioni e gli assegni familiari, le famiglie pagheranno meno tasse: se ne

campo del lavoro precario con la stabilizzazione nel settore della scuola e la novità del Fondo della pubblica amministrazione. È un primo segnale

Ci hanno accusato di essere contrari alla sistemazione e allo sviluppo dei porti, che è un tema strategico nel nostro Paese. Noi vogliamo che questo sistema venga sviluppato, ma nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e con le valutazioni di impatto al tema delle rottamazioni, si tratta di una norma che non abbiamo voluto noi, ma che abbiamo predisposto per garantire ai Sindaci la possibilità di intervenire per migliorare la qualità e la vivibilità delle città. Eppure, signor Presidente, mi rivolgo direttamente al Governo ci sono due temi di grande sofferenza per i Verdi e per tutto il nostro Gruppo. Gruppo. Mi riferisco anzitutto alla questione del CIP 6, che, tradotto, significa che gli incentivi, che dovrebbero essere assegnati alle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, saranno assegnati anche alle cosiddette fonti assimilabili. significa che vengono bruciate delle sostanze che producono schifezze in atmosfera e che, in più, ricevono gli incentivi. Questi incentivi sono pagati dai contribuenti. Questa è una vergogna che deve finire. questa è una vergogna che deve finire! Il Parlamento si deve far carico di questo tema. Noi lo abbiamo affrontato e abbiamo raggiunto un accordo nella maggioranza e con il Governo. Prendiamo atto

solo con l'intesa di una parte della maggioranza. Se si fanno operazioni di questo tipo, bisogna avere il consenso di tutta la maggioranza. C'è poi un problema di merito

di sani regolamenti che attengono alla rigorosa procedura per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per la loro gestione.

Noi vogliamo combattere l'evasione. Combattere l'evasione, avere maggior gettito dal punto di vista della lotta all'evasione fiscale, significa aumentare le tasse? Io credo di no.

capire che la nostra gente ha bisogno di un futuro sereno, di vivibilità, di salari adeguati, di diritti, di salute, di cibi sani per i propri figli. Per dare queste risposte, dobbiamo

onesta che lavora, gente leale, darà la fiducia a questo Governo. Ma noi chiediamo al Governo di avere più fiducia in tutta la sua maggioranza. Se ci sarà questo rapporto, noi ci saremo e ci saremo fino in fondo, con la lealtà che contraddistingue il nostro lavoro. *(Applausi

che il Governo chiede al Parlamento in sei mesi di vita: un record, che testimonia, da un lato, la tendenza antidemocratica che lo contraddistingue e, dall'altro, la intrinseca debolezza da cui è attanagliato. Troppi, infatti, i rischi per affrontare un dibattito in Aula, troppe le contraddizioni all'interno della maggioranza per garantire un indirizzo coeso sugli emendamenti, e troppo poca forse la confidenza che i senatori a vita, fondamentali per la tenuta della maggioranza stessa, potessero sopportare il tedio, la fatica della discussione in Aula sulla legge finanziaria. Oggi si consumerà l'ennesimo vuoto rito, grazie al quale il Governo otterrà la fiducia del Senato. Sono infatti stati tutti precettati coloro che garantiscono un numero di voti irraggiungibile per l'opposizione, a partire dai già citati senatori a vita. Ma a nessuno credo sfugga l'atmosfera un po' surreale che qui stasera si respira. Sicuramente aleggiano in quest'Aula le parole dei rettori, che ieri hanno dichiarato, a testimonianza del loro profondissimo disagio: Ministri non vi vogliamo, non fatevi più vedere nelle università. A tale proposito, sarebbe interessante conoscere il parere della senatrice Levi-Montalcini, visto che ha sempre dichiarato che non avrebbe votato la finanziaria, se essa non fosse stata soddisfacente per la ricerca. ricerca. In campagna elettorale, non più tardi del 15 marzo 2006, il futuro presidente Prodi rilasciava dichiarazioni di questa natura: «È possibile organizzare un po' di felicità per noi». Come è amaramente diversa la realtà! Fantasie sognate dal capo di un Governo che sta dando di sé - sono parole di Eugenio Scalfari, non mie - un'immagine scomposta, sciancata, mediocre. Alla prova dei fatti, la legge finanziaria ha rivelato la sua vera natura: una legge livorosa, vendicativa, fatta - secondo voi - contro i ricchi, che finalmente avrebbero pianto. Ma chi sono per voi i ricchi? Quelli che hanno un patrimonio superiore a 180.000 euro, disse il non ancora presidente Bertinotti in campagna elettorale, cioè tutti coloro che hanno un appartamento in città e coloro che percepiscono un reddito superiore a 1.350 euro, come dice questo testo, cioè i ceti produttivi, i lavoratori, gli artigiani, i professionisti, i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi, che si sono ribellati, sono scesi in piazza a protestare, a gridare tutta la loro rabbia contro questa finanziaria ingiusta, vessatoria e penalizzante verso il Nord, che - non dimentichiamolo - produce la maggior parte del prodotto interno lordo del Paese. Ma, colleghi della sinistra, non vi sorge il dubbio che vi sia qualcosa che non va, qualcosa di sbagliato o di storto in questa legge? Plaudono adesso la grande industria, i massimi vertici sindacali - non i lavoratori, si badi bene, come le recenti vicende di Mirafiori hanno dimostrato - le grandi banche, mentre non la sopportano, al punto da scendere in piazza, i tassisti, gli artigiani, i commercianti, i pompieri, gli agenti di polizia, i liberi professionisti, i sindaci, i pensionati, il mondo della scuola, insomma quasi tutta la società civile, per usare un termine a voi della sinistra molto caro. E poi vi illudete che i fischi siano organizzati.

avete aumentato le tariffe dei treni, il bollo per auto e moto, i telefoni, le spese mediche, i parametri degli studi di settore, le tasse di successione, il canone RAI, pagato soprattutto dai meno abbienti, avete scippato i conti correnti dei morti nonché il TFR ai lavoratori.

Questa è la risposta che ha dato il Presidente del Consiglio. Gli italiani sono matti e non capiscono quanta è buona questa finanziaria. Per questo protestano, anzi non capiscono la natura salvifica e quasi catartica di questa manovra.

A tal proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare che non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale». Ebbene, signor presidente Ciampi, lei ci ha appena detto che voterà in maniera convinta un mostro di un articolo con 1.365 commi. La coerenza, purtroppo, va sacrificata alla ragione politica e di questo ci dispiace profondamente. Sono le tristi necessità della politica. Colleghi, questa finanziaria è in linea con la politica di questi sei mesi legata ad un Governo che vuole un mondo a rovescio. Avete liberato i criminali con l'indulto e criminalizzate gli onesti cittadini sottoponendoli ad asfissianti indagini da grande fratello, ritenendoli tutti pericolosi evasori. Lasciate liberi, con il provvedimento del ministro Turco, i nostri giovani di bruciarsi il cervello con gli spinelli, ma per i luoghi in cui i nostri ragazzi si formano, la scuola e l'università, date meno soldi e, di più, li istigate al gioco d'azzardo ampliando notevolmente l'offerta di giochi, anche in questo caso per lucrare soldi. Ritenete i lavoratori autonomi italiani degli evasori di cui non fidarsi e da controllare strettamente in ogni loro manifestazione, anche privata, e consentite agli extracomunitari di ottenere detrazioni, attraverso la semplice produzione di documentazione del Paese d'origine, praticamente impossibile da controllare. Siete contro la famiglia che gli italiani vogliono, quella che genera i figli attraverso l'unione tra uomo e donna, ma volete quella omosessuale e vi accingete a portare avanti i Pacs, che prevedono anche la famiglia omosessuale. Un mondo a rovescio: un mondo a gambe all'aria, che però non può stare in piedi! Qui voi cercate la fiducia e qui, nel chiuso del Palazzo, la otterrete, ma fuori, nel Paese che vive e che produce, l'avete già irrimediabilmente persa: non vi crede più nessuno. Il Paese vi ha sfiduciato, vi hanno sfiduciato le agenzie di *rating*. Il più importante quotidiano economico internazionale ha definito il nostro Ministro del tesoro «il più incompetente d'Europa». Avete fallito: non siete più credibili. E allora, stasera, non soltanto a nome della Lega Nord dichiaro il voto contrario, ma credo anche a nome della stragrande maggioranza del Paese. E mando a dire a Prodi, che qui non c'è e che si è rifiutato di seguire questo dibattito: in democrazia, un Governo quando non ha più la fiducia degli elettori si dimette e va a casa; vada a casa, faccio un regalo agli italiani per Natale, Presidente!

*(UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questa è la più brutta finanziaria per il bilancio delle famiglie italiane degli ultimi anni, nonostante sia la finanziaria della CGIL, dei Verdi, di Bertinotti e Diliberto. Alla fine del 2007 saremo tutti più poveri, soprattutto chi è già povero, perché l'Italia sarà più povera, come già hanno giudicato le agenzie di *rating*. Il disagio sociale si è già manifestato con centinaia di manifestazioni di protesta. Non passa giorno che a Roma non ci sia un corteo spontaneo contro il Governo Prodi. Il disagio politico è evidente dentro la maggioranza e a maggior ragione è espresso dall'opposizione. Il 2 dicembre scorso l'UDC a Palermo e il resto della Casa della Libertà a Roma hanno fatto sentire forte e chiaro il proprio no a questa finanziaria e a questo Governo. Il nostro no, come ha spiegato Casini, non è pregiudiziale: è un no ragionato, un no per il bene dell'Italia. Chi protesta e dissente è la stessa Italia che ha votato Prodi: Sindaci di centro-sinistra, Ministri, Sottosegretari, *leader* di maggioranza ogni giorno hanno qualcosa da dire contro questa finanziaria. Prodi ha detto che siamo impazziti tutti. Probabilmente è vero, perché è una finanziaria da far diventare pazzi solo a leggerla: 1.365 commi. Mai successo nella storia del Parlamento! Anche le cifre faranno impazzire gli italiani: 40 miliardi di euro è il valore della manovra. Il bollettino economico della Banca d'Italia di qualche settimana fa ha fornito i seguenti dati: 24 miliardi di euro è il peso delle maggiori entrate; 13 miliardi di euro è il peso della maggiore spesa. Più entrate significa più tasse per gli italiani; più spesa significa mantenere ancora privilegi, sprechi e carrozzoni inutili. La vostra esperienza è fallita quando avete nominato 103 uomini di Governo e oggi confermate agli italiani che siete dei pessimi spendaccioni. Il presidente Ciampi si era chiesto, qualche mese fa, se questa finanziaria avesse una missione, se avesse cioè uno scopo, un fine. Prodi ha risposto che gli obiettivi erano: risanamento, sviluppo ed equità sociale. In questo maxiemendamento non troviamo misure a favore di simili obiettivi. Il vice ministro Visco, qualche giorno fa, ha dimostrato che rispetto al 2005 lo Stato ha incassato maggiori entrate per oltre 29 miliardi di euro. Il ministro Padoa‑Schioppa ha dichiarato che, per riportare il *deficit* sotto il 3 per cento, bastavano 15 miliardi di euro. Anche un bambino delle elementari capirebbe che bastavano le maggiori entrate registrate, proiettate al 2007, per evitare nuove e maggiori tasse. Invece no. Da quando vi siete insediati avete messo solo tasse a chi lavora e, con la scusa dell'evasione fiscale, che è un furto (come dice il presidente Casini), avete messo sotto sorveglianza ogni nostra azione economica, anziché applicare il contrasto di interessi. Queste tasse non servono allo sviluppo, ma per pagare spese localistiche settoriali e clientelari, come dimostra il maxiemendamento, che indica anche il nome del proponente. Il vizio di fondo, la debolezza politica di questa maggioranza sta nel ricatto permanente di personaggi senza scrupoli, che, vostri alleati, fanno pesare il loro voto determinante sulle spalle dello Stato, della collettività e degli italiani. Un esempio per tutti: il comma 1346, un regalo ai predatori dello Stato. In tutti i campi del lavoro umano, chi sbaglia paga. Qui, dipendenti pubblici ed amministratori, che sono sotto processo per danni allo Stato e agli enti pubblici, vengono amnistiati. Molti di voi dicono che avete subito un ricatto. Il senatore Salvi, addirittura, indica un potente Ministro di questo Governo quale beneficiario della norma, perché inquisito per danni patrimoniali quando era sindaco di Roma. Forse si tratta di un colpo di spugna? Oppure è una legge *ad personam*?

di questo o quel partito, di questo o quell'altro schieramento. Siamo contro questa finanziaria anche perché non ci è piaciuto il ricatto politico, la vendetta odiosa contro la Sicilia di Cuffaro. Nemmeno Camilleri ha capito la cancellazione del ponte sullo Stretto di Messina e la restituzione dei finanziamenti all'Unione Europea. A parte le società che gestiscono i traghetti, non c'è siciliano che abbia capito perché deve rimanere staccato dall'Europa. Non hanno capito decine di ricercatori, e nemmeno Dario Fo e Franca Rame (che ringrazio), perché avete prima cancellato e poi tagliato i fondi per il Centro di ricerca sulle biotecnologie di Carini in Sicilia. Non abbiamo capito perché avete tagliato 700 milioni di euro al bilancio della Sicilia, con un credito di imposta sulle attività produttive che paga la stessa Sicilia e non lo Stato. Un'ingiustizia che l'UDC non ha accettato e cui si opporrà in tutti i modi e con tutte le proprie forze, insieme ai siciliani. Negli ultimi dieci anni, la ricchezza del Paese (cioè il PIL) in Italia è cresciuta del 12,7 per cento, nell'Europa dell'euro del 20,5 per cento, negli Stati Uniti del 33,3 per cento. Nel mercato globale l'Italia ha quindi una velocità che è quasi la metà di quella europea e quasi un terzo di quella degli Stati Uniti.

quelle italiane solo del 20 per cento. Mentre gli altri corrono, noi stiamo quasi fermi. Quote di mercato estero italiano sono state occupate dai Paesi emergenti: Cina, India, Brasile, Vietnam, Corea del Sud, Sudafrica. Se è vero che un cinese lavora 3.600 ore, rispetto alle 1.700 di un italiano, e ha una retribuzione 20 volte inferiore, significa che la sfida non è sul costo del lavoro o sul prezzo, ma sulla qualità dei prodotti e, quindi, sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca. L'Italia deve investire sulle intelligenze, l'Italia deve investire sulla scuola, sulle università, sui giovani, sul futuro. Il sistema produttivo italiano deve riconvertirsi in fretta e adeguarsi alla domanda mondiale. Basta con i privilegi corporativi, con le rendite di posizione, con la difesa dei monopoli pubblici e privati. Dobbiamo aprire un'altra stagione politica, fondata sul confronto e non sullo scontro. Noi dell'UDC abbiamo iniziato un autonomo cammino politico, perché possa essere premiata, o almeno non punita, quell'Italia che studia, si sacrifica, lavora, intraprende e rischia in proprio, affinché l'orgoglio italiano torni a primeggiare nel mondo. In questa finanziaria abbiamo giudicato negativamente l'esproprio del TFR dei lavoratori, trattenuto dalle aziende per destinarlo all'INPS al fine di finanziare infrastrutture, così come abbiamo denunciato l'imbroglio della riduzione del cuneo fiscale. Prodi aveva promesso cinque punti nei primi 100 giorni, con vantaggi alle imprese e ai lavoratori dipendenti: niente ai lavoratori dipendenti, solo sgravi fiscali sull'IRAP per le imprese. Invece di abbassare i costi di produzione e sostenere sui mercati esteri le aziende più dinamiche, si abbassa solo il costo del lavoro, allungando l'agonia di qualche grande azienda che non riesce a stare sul mercato globale. Questa finanziaria non solo non crea sviluppo, ma è anche iniqua socialmente. Esiste un principio da rispettare in economia e in politica: la ricchezza prima si crea e poi si può distribuire: se distribuiamo solo quella che c'è, per cui anche i ricchi piangono, alla fine del 2007 i poveri si dispereranno. La riforma dell'IRPEF e la propaganda del Governo sostengono che a guadagnarci sono i redditi sotto i 20.000 euro,

anche addizionali sull'IRPEF dei Comuni e delle Regioni, l'imposta ICI sulla prima casa, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa sul gasolio con l'aumento dell'accisa regionale, le tasse di circolazione per auto e motocicli, la tassa sulla salute con i *tickets* sulla sanità, oltre all'imposta di scopo, all'aumento sui diritti di imbarco, sui visti d'ingresso e perfino una tassa di un centesimo su ogni bottiglia di acqua minerale con la quale, se ci fosse stata insieme quella sul pane, ci avreste ridotto a pane ed acqua. Aumentano inoltre, e concludo, Presidente, le tariffe sul trasporto pubblico, la luce, l'acqua, il gas e, è notizia di oggi, anche il canone TV. Avremmo voluto confrontarci con questa maggioranza, se non si fosse chiusa e blindata sul DPEF di luglio, cioè su quello che propone di rivedere, attraverso le liberalizzazioni, le nuove tariffe dei servizi pubblici locali, di modernizzare le infrastrutture e di avere un Paese più moderno e più nuovo. sperando di avere un altro Governo e un'altra maggioranza.

Invece dei soliti titoli, l'intera prima pagina conteneva i nomi dei 246 morti sul lavoro nei primi mesi del 2006 nel solo settore dell'edilizia: morti perché lavoravano senza protezione, schiavi uccisi da una strage liberista in Italia, guardate, non nelle zone franche cinesi o nelle miniere ucraine o nelle fabbriche del sudore del Guatemala o del Nicaragua. Andrea, Luigi, Mario, Rosario, Nexhat, Mohammed: ci vorrebbero tante e tante prime pagine con le liste dei nomi dei tanti torturati, dei tanti morti di fame e di guerra. Noi vorremmo dare un po' di voce alta a quanti stanno in basso, a quei milioni di italiani ed italiane che vivono in un cono d'ombra, in un mondo sommerso. Forse il cavalier Berlusconi considera comunista questa finanziaria perché, come maggioranza, ci siamo battuti per l'assunzione di 300 nuovi ispettori del lavoro, affinché si salvi qualche ragazzo che ogni giorno muore schiacciato da un carrello, mentre lavora per pochi soldi. Certo, a Berlusconi appare scandaloso che questa finanziaria invece di condoni e pene agli evasori tenti, per quanto timidamente, di cambiare impianto, mutare impostazione, iniziare un percorso di redistribuzione ed equità sociale, di nominare perlomeno la narrazione di vita quotidiana del nostro popolo. No, non è la finanziaria che avremmo voluto: vi sono elementi di sofferenza nella scuola, nella ricerca, nell'università, nei fondi delle energie rinnovabili erogate per gli inceneritori e per i petrolieri, ma vi è, comunque, un mutamento di paradigma, di priorità, di referenti sociali. Un primo passo nella direzione giusta. E le nostre compagne e i nostri compagni, che ringrazio, pur nell'articolazione delle loro posizioni, hanno svolto un ruolo importante nelle Commissioni per accrescere il suo tratto sociale. Qual è infatti la concezione delle destre? Una coincidenza tra valori e interessi proprietari. Da un lato, lo Stato etico e patriarcale contro le donne, giustizialista, proibizionista, razzista, dall'altro, la negazione alla radice dello Stato sociale, inteso come rapporto tra individuo e contratto sociale. Stiamo parlando di saperi, di culture, ma anche di infrastrutture, di treni per i pendolari, di acque, dei beni comuni come valore d'uso collettivo, non come merce privatizzata. Stiamo parlando di sanità. È stato importante abolire l'odioso *tickets* sul pronto soccorso. soccorso. La politica vera, per non essere una chiacchiera autoreferenziale o una accademia elitaria e separata, deve saper riconoscere i soggetti sociali, ha bisogno della materialità dei corpi, delle vite.

che era presente nella famosa assemblea della FIAT Mirafiori, quell'assemblea che ha posto a noi domande alle quali sentiamo il dovere di rispondere: «Sono entrata in FIAT nel 1979» - dice Caterina - «Ero, giovedì, all'assemblea sindacale delle carrozzerie e ho visto alcune mie compagne, che, come me, guadagnano 1.100 euro al mese, urlare perché si sono ammalate di tendinite. Qui, sapete, in fabbrica, siamo tutti un po' malmessi. Chi ha la periartrite, chi ha il mal di schiena, chi ha problemi al tunnel carpale. I turni poi in fabbrica ti sballano tutta la vita. Per anni ed anni io e mio marito ci siamo incontrati soltanto la domenica. Mia figlia non l'ho vista crescere. Sono andata e venuta a settimane alterne e il tempo è passato, è passato». Caterina e i milioni di Caterina vanno rimesse al centro della nostra politica. Caterina ci dice che negli ultimi 25 anni le risorse destinate ai salari sono scese dal 70 al 48 per cento, che vi è stata una crescita enorme delle disuguaglianze sociali. Allora occorre cominciare ad operare politiche redistributive, di risarcimento sociale. Esse devono rappresentare il cuore della nostra politica economica. Non può ripartire l'economia se non vi è l'innalzamento della quota della ricchezza sociale prodotta, da destinare ai redditi da lavoro. Ci siamo impegnati in questa finanziaria per cominciare a dare diritti e stabilizzazione ai precari. I precari della scuola saranno stabilizzati in 250.000; migliaia e migliaia di precari della pubblica amministrazione saranno stabilizzati. Certo, è ancora poco, è solo l'inizio. Noi vogliamo che la lotta alla precarietà diventi una carta d'identità del Governo, come oggi lo è la lotta all'evasione fiscale. La precarietà, infatti, non è soltanto un aspetto del mercato del lavoro, è privazione di senso, incertezza del futuro. I nostri figli e i nostri nipoti ce lo dicono con sofferenza, di fronte ad un lavoro che è nomade, che ora c'è e ora non c'è, che appare e poi scompare. Di fronte ad un lavoro nomade, sociale; è un dato perfino antropologico: il lavoro precario genera rapporti precari di tempo, di spazio, di relazioni, di amori, di vite. Diceva un volantino dei nostri giovani precari che ho letto qualche settimana fa: la precarietà ha sostituito il diritto al lavoro con il dovere di dimostrarsi occupabili ovvero devi essere più conveniente del tuo amico sul mercato, più disposto ad accettare restrizione di salario e diritti. É vero ed è tremendo: chi inneggia alla precarietà ci pensi! Essa è l'orizzonte della solitudine competitiva, una competizione inumana, nella quale scompare qualsiasi idea di legame sociale, di spazio pubblico e condiviso dei diritti, di comunità democratica, di sindacato persino. Questo volevamo dire quando siamo andati in piazza il 4 novembre all'interno dei movimenti di lotta contro la precarietà, così come lo siamo stati in questi giorni con i pensionati, gli universitari, i ricercatori, le comunità in lotta contro la TAV, il MOSE, il Ponte sullo Stretto che finalmente questa finanziaria cancella. Abbiamo fatto scandalo per i benpensanti. Siamo stati in piazza con i precari, noi parlamentari, le donne e gli uomini di Governo di Rifondazione Comunista. Sia chiaro: io penso che sarebbe stato scandaloso se non ci fossimo andati in quelle piazze. Ma chi diavolo ha mai detto che se sei in maggioranza o al Governo devi separarti dalla lotta e dalla condizione sociale? Per noi il Governo è un mezzo, non è un fine. Le donne e gli uomini di Rifondazione Comunista non pensano che la politica si faccia solo nelle Aule parlamentari. Siamo responsabili e quindi siamo disobbedienti. Siamo qui in queste Aule, partigiani convinti e determinati di questa maggioranza, di questo Governo, che vive nella forza del suo programma. Non c'è una fase 1 ed una fase 2. Ha ragione il presidente Prodi. C'è solo l'Unione, il suo programma e bisogna realizzarlo perché è il nostro popolo, quello che ci ha voluto al Governo, che è in credito, che vuole più democrazia, più socialità, più convivialità, più ascolto vorrei dire. E noi vogliamo ascoltare. Siamo qui, ma per questo saremo anche martedì ai cancelli di Mirafiori, saremo nelle case occupate per rivendicare il diritto all'abitare. Saremo, come ha fatto Haidi Giuliani nei giorni scorsi, nei centri di permanenza temporanea, vere e proprie galere etniche dove sono rinchiusi ingiustamente sorelle e fratelli emigranti. È il nostro contributo a questa maggioranza. Ma non è un azzardo. Siamo convinti che il Governo Prodi avrà ampi consensi se saprà distanziarsi sempre più dal berlusconismo, suscitando partecipazione, protagonismo, anche conflitto sociale, del quale non dobbiamo aver paura perché è il sale della democrazia democrazia ed è una necessità per costruire più ampi rapporti di forze e più consenso a livello sociale. Se il popolo dell'Unione si dividesse, ma se soprattutto si rinchiudesse in una cupa ed amara delusione o in una delega rassegnata a noi**,** al Governo sarebbe la sconfitta della politica, sarebbe la vittoria dell'antipolitica. Ma è proprio questa convinzione, questo amore per il nostro popolo che esprime bisogni e che pretende da noi soluzioni, che ci dà forza e fiducia. E noi dobbiamo realizzare ogni giorno orizzonti di libertà e percorsi di uguaglianza. Lo sappiamo e, soprattutto, per il nostro popolo lo vogliamo.

Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, voglio prima di tutto ringraziare il presidente Marini per l'equilibrio dimostrato, per aver respinto il tentativo del Governo di far rimediare al Presidente del Senato alle brutte figure del Governo stesso ed un grazie al presidente della Commissione bilancio, senatore Morando,

parte degli italiani. Perché? La riduzione del cuneo fiscale è ritenuta dalla maggioranza del Paese insufficiente; gli aumenti delle tasse per i redditi più elevati sono parsi inutilmente punitivi; il passaggio all'INPS di 65 miliardi sottratti al TFR è stato accolto come un esproprio; le nuove tasse che gli enti locali finiranno con l'essere obbligati ad introdurre danno la sensazione che il Governo preferisca lasciare ad altri la responsabilità di imporre nuove gabelle; l'operosità del Paese viene ignorata, i professionisti considerati solo come evasori fiscali. Queste note non sono mie, ma le leggiamo su autorevoli giornali che hanno appoggiato la campagna elettorale del centro-sinistra. Questa finanziaria è stata criticata e bocciata da tutti i più grandi organismi internazionali, dall'OCSE alle Agenzie di *rating,* dal Fondo monetario internazionale alla Banca d'Italia, dalla Confindustria e, dopo le proteste ed i fischi di Mirafiori, anche dai sindacati confederali. I rettori delle università

la collega Levi-Montalcini, tanto sensibile a queste problematiche. Professionisti, farmacisti, lavoratori autonomi, uomini di cultura, lavoratori dipendenti, pensionati scendono in piazza uniti per protestare. una finanziaria dove vengono introdotte norme clientelari accanto alle quali c'è scritto il nome ed il cognome dei proponenti, minitasse sulle bottiglie dell'acqua minerale. Sui *manager* di Stato viene stabilito un tetto retributivo, ma subito dopo viene introdotta una norma con scritto «Il Governo può derogare». Fondo precari: viene istituito un fondo di appena 5 milioni, che servirà a stabilizzare 200, 250 precari, anziché 350.000 promessi. Aumentano i pedaggi autostradali, ma non si sa di quanto. Vengono tagliate del 5 per cento alcune spese per le strutture della Polizia. Per la campagna di educazione dei giovani, finalizzata alla conoscenza dei rischi derivanti dal gioco, vengono stanziati, dico, vengono stanziati, 100.000 euro; insufficienti anche a pubblicare un solo manifesto. Forse si doveva dare uno stipendio ad un amico degli amici. *(Applausi dai Una manovra, quindi, senza padri; uscita dal Consiglio dei ministri il 30 settembre era già cambiata al suo arrivo alla Camera: 20 metri di tragitto. Una manovra che è stata modificata dal Governo oltre 100 volte, con i parlamentari della maggioranza messi nelle condizioni di non poter incidere. Una manovra che porta in sé un aspetto politico di grande rilevanza, la sconfitta dei riformisti, che, pur essendo maggioranza, in cambio della loro permanenza a Palazzo Chigi, sono rimasti a fare le comparse: zitti e mosca! *(Applausi l'aspetto politico più chiaro che viene fuori dalla manovra finanziaria: due terzi dei parlamentari dell'Unione sottomessi alla restante parte rappresentano il fatto politico più significativo. E quando ieri l'onorevole Fassino, segretario del partito di maggioranza relativa della coalizione, ha fatto una diagnosi coraggiosa al suo partito di questi sei mesi di Governo, ammettendo il fallimento dovuto alla dovuto alla «cattiva dialettica tra l'ala riformista e quella radicale della maggioranza» e indicando come terapia il cambio di passo o addirittura di rotta, stato zittito e trattato con sufficienza dal Presidente del Consiglio. E non vale il tentativo di nascondersi dietro le parole, perché è chiaro a tutti che Prodi risponde no a Fassino. Non ci può essere quindi cambio di passo al punto in cui siamo arrivati, bensì solo un cambio di Governo e soprattutto un cambio di Presidente del Consiglio. È fin troppo facile la conclusione: mandiamo a casa Prodi. Prodi è l'unico, purtroppo, che non ha notato quanto gli accade intorno. Il 2 dicembre, a Roma, hanno manifestato 2 milioni di cittadini, merito degli organizzatori certamente, ma il principale merito va al Presidente del Consiglio, che con i suoi provvedimenti ha scatenato l'ira degli italiani. e FI)*. Lei, Presidente del Consiglio, passando da una *gaffe* all'altra, fino a pochi giorni fa ha tra l'altro detto: «Il Paese è impazzito...», fino ad arrivare ieri a dichiarare testualmente: «Rifarei la finanziaria identica, ma in modo diverso». Come si fa a fare una cosa identica e diversa allo stesso tempo ce lo spiegherà quando avrà un po' di tempo. Lei, signor Presidente del Consiglio, è ormai in rotta di collisione con se stesso, con il Paese e con la lingua italiana, e, mi creda, sono convinto che sia entrato in rotta di collisione anche con la parte moderata della sua maggioranza. L'ultima prova è arrivata ieri, quando con una sola battuta ha detto: «Non parliamo di fase 2», snobbando la relazione politica svolta dall'onorevole Fassino al suo partito e la richiesta fatta dall'onorevole Rutelli. Per il bene del Paese è opportuno che si faccia da parte. vedremo insieme, maggioranza e opposizione, quale sarà la soluzione migliore per l'Italia e per i cittadini, se riandare al voto immediato, cosa che auspico, o se varare un Governo breve e transitorio, che prenda pochi provvedimenti sul piano economico e istituzionale

Direbbe Leo Longanesi, giornalista, scrittore, dissacratore di usi e costumi: cosa voglia Prodi si sa. Vuole esistere e durare; per esistere egli non ha trovato di meglio che fare l'uomo di sinistra, come altri fanno il notaio o l'avvocato; ormai si è così abituato e convinto di essere sempre stato di sinistra, si è fatto un repertorio di frasi che non mutano, se le ripete e gli sembrano nuove, così tira avanti tra un voto di fiducia e un altro, ma tutto ciò è soltanto un equivoco, una finzione, un pretesto. Il suo essere di sinistra non ha forma, i suoi programmi politici sono impostati soltanto sul togliere e sul distribuire e fa finta di non accorgersi che la sinistra, padrona della maggioranza, lavora, non con l'obiettivo di far stare tutti meglio, ma di livellarci al peggio. Altra è la filosofia politica che ci anima. La destra si ispira a principi di sussidiarietà e vede lo Stato come elemento equilibratore dei processi di concorrenza e competizione; lo Stato come equilibratore e arbitro, non destinato ad intervenire ovunque e comunque. In sostanza, vogliamo riaffermare nei fatti il primato della politica che non porti a truccare le carte, come avete fatto, nascondendo 37-38 miliardi. il Presidente del Consiglio si interroga sui fischi, si è convinto che qualcuno organizzi la protesta contro di lui, riducendo a dei teppistelli chi va a fischiarlo. un brutto passaggio: quando in piazza va la sinistra, sono cittadini che democraticamente protestano; quando ci vanno altri, ricevono l'epiteto di teppistelli. Attenzione, è vero, dietro i fischi c'è un grande organizzatore, un uomo bravissimo che è capace di indurre tutti alla protesta e quindi ai fischi: è lei stesso, signor Presidente, con le sue decisioni, con i suoi provvedimenti e, soprattutto, è lei quando spiega perché sono state varate certe norme. «Tutti avversano la finanziaria?» - si chiede e lei risponde - «Bene, bene, bene!» Altro che fischi, presto arriveranno anche gli ortaggi.

analogo ringraziamento al Presidente del Consiglio, il quale ha sentito il dovere e il piacere di ascoltare il suo Ministro, ma non un analogo rispetto nei confronti di questo Parlamento per i nostri interventi; eravamo abituati a ben altro.

un'Italia con una pressione fiscale al 41,6 per cento, la minore in assoluto degli ultimi decenni, il tasso di disoccupazione al 7 per cento, un'inflazione sotto il 2 per cento, nessun buco nei conti, come è accertato dalla Banca d'Italia, uno stanziamento, accertato dal CIPE, di ben 50 miliardi per opere infrastrutturali, maggiori entrate per 34 miliardi, confermate vice ministro Visco, una crescita del PIL del Paese in linea con quella europea dell'1,9 per cento: questa è l'Italia che il Governo Berlusconi ha lasciato in eredità. Ci troviamo ad assistere ad una finanziaria che balla da due mesi, di un'entità variabile: variano le tasse, le controtasse, le diminuzioni;

una finanziaria basata su maggiori entrate e su totale assenza di tagli strutturali; una finanziaria che aumenterà la pressione fiscale fino a più del 44 una finanziaria che non piace nemmeno allo stesso Governo che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, ha visto marciare sottosegretari del Governo contro lo stesso Prodi in piazza. una finanziaria bocciata all'estero, dall'OCSE, dalle agenzie di *rating*, da 30 associazioni di categoria che sono scese in piazza a protestare; da tutti i professionisti e da tutti i produttori di reddito. Ma è un disegno di legge finanziaria che non piace allo stesso Governo. Mi limito a denunciare alcune battute di alcuni illustri autorevoli Ministri di questo Governo. Ferrero: su povertà non c'è quasi nulla; D'Alema: una manovra indigesta a causa dei nostri errori; Amato: anch'io posso collocarmi tra gli scontenti di questa manovra finanziaria; Rutelli: i conti sulla cultura non tornano; Mussi: migliorare la finanziaria in Senato; la collega Finocchiaro, oggi, su «La Stampa»: tutti abbiamo visto instabilità decisionale venire dal Governo.

pesa la difficoltà di promuovere e realizzare una condivisione fondata su un riconoscimento del ruolo della società e dei suoi soggetti. Egli ha ragione, ma ha sbagliato nel rapporto con i soggetti della società, perché ha attivato un odio

Ecco perché ha sbagliato: ha modificato le norme professionali attraverso una decretazione d'urgenza, senza alcuna concertazione con le categorie professionali.

Semplicissimo. E invece no. Cosa si è fatto? Si è messa su una maximanovra: tassazione del Paese per redistribuire la ricchezza. E come mai a Mirafiori gli operai hanno contestato i sindacati? Voi ve lo chiedete? Noi ce lo chiediamo.

i pedaggi autostradali aumenteranno; pagheranno di più per i trasporti pubblici; pagheranno i *ticket* sanitari sulle ricette specialistiche e sul pronto soccorso; aumenteranno le tasse locali emesse dai Comuni e dalle Regioni; aumenterà l'ICI; aumenterà la tassazione sui risparmi, il gasolio da riscaldamento, l'acqua minerale, il canone RAI,

al Fondo per le aree sottosviluppate e, nello stesso tempo, si pensa a dare dei contributi - udite, udite - ai raccoglitori di miele nei boschi. Questa è la manovra finanziaria del Governo Prodi. Abbiamo lasciato, con il nostro Governo, una politica fiscale che ha dato i suoi frutti; esso è sotto gli occhi di tutti:

Siamo stati invitati a confrontarci da autorevoli esponenti della maggioranza in Senato. Ci è stato detto: vogliamo ascoltare le vostre proposte. confrontiamoci, siamo aperti al dialogo. Ci siamo presentati in pompa magna davanti alle televisioni e ai giornalisti, abbiamo manifestato le nostre proposte, abbiamo affermato una cosa semplice: vi abbiamo lasciato un *surplus* di entrate fiscali? È conclamato?

Ci è stato risposto che non era possibile; che se ne sarebbe parlato da gennaio e quindi nulla si poteva cambiare. Così nemmeno quella norma assurda e inverosimile, secondo la quale il TFR, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori, da posta debitoria all'interno delle imprese, diventa in questa manovra finanziaria un'entrata per lo Stato. Ancora vorremmo capire come.

Gruppo FI)*. Questa è una finanziaria contro lo sviluppo e non per lo sviluppo. Avevamo chiesto maggiori risorse per le infrastrutture e la sicurezza. Apprendiamo invece che nel maxiemendamento si realizzano tagli alle spese correnti delle forze dell'ordine e si prevede la possibilità di chiusura di questure e prefetture.

a concludere - lo scandalo del comma 1346, cioè la sanatoria sui reati contabili contro la pubblica amministrazione.

Signor Ministro dell'economia, signor Ministro della giustizia, Sottosegretari presenti, il testo sul quale il Governo ha posto il voto di fiducia reca netto il segno del contributo del Gruppo dell'Ulivo e degli altri Gruppi dell'Unione al Senato su questioni di merito di grande rilievo politico, ma c'è un altro segno politico essenziale. Mi riferisco alla coesione e alla reciproca, solidale partecipazione con la quale le forze dell'Unione hanno lavorato qui, evidente nella rappresentazione pubblica e nella lettura che ne hanno fatto gli osservatori politici e mediatici: un segnale di svolta rispetto al clima delle settimane precedenti. I due risultati, quello di merito e quello politico, non sono un'accidentalità. Sono costati molto lavoro, molta intelligenza politica e un grande senso di responsabilità e non sono classificabili sotto la voce «tributi al Governo»; nascono da un'autonoma decisione politica e hanno avuto un riferimento e un fine principale.

l'ansia delle famiglie con un reddito basso e, per questo, abbiamo provveduto alle nuove misure in materia di assegni famigliari e detrazioni IRPEF. Abbiamo guardato al senso di devastante precarietà dei ragazzi e delle ragazze italiane, ma anche di uomini e donne, di fronte all'assenza di diritti e di prospettive di futuro. Per questo, siamo intervenuti con le misure sul lavoro precario: sulla stabilizzazione e sui diritti del lavoro precario e sulla contribuzione degli apprendisti. Vorrei ancora dire che abbiamo guardato ad un altro bisogno, quello di autonomia, al primo desidero di chi voglia rendersi autonomo, al desidero di avere una casa, di poter avere una famiglia, con il primo con il primo investimento dopo 20 anni sull'edilizia residenziale pubblica. Ricordo poi le questioni del *ticket* sanitario per rispondere al bisogno e alla sicurezza sulla salute e, ancora, gli interventi che abbiamo fatto sui Comuni nella consapevolezza che qui si costruiscono la prima cittadinanza e i primi diritti dei cittadini. Abbiamo aggredito, per la prima volta, la questione dei costi della politica. Colleghi, guardate in controluce: queste misure rivelano altro che una finanziaria senz'anima. In queste misure c'è un'idea dell'Italia, ed è l'Italia seria e rigorosa, che in quest'Aula, poco fa, il ministro Padoa-Schioppa ha dato con la sua relazione e che - lasciatemelo dire - tante volte nelle Aule della Camera e del Senato ha dato il ministro per l'economia Carlo Azeglio Ciampi. Lo voglio ricordare e lo voglio dire così: è l'Italia del dovere pubblico prima di essere l'Italia dei poteri. Ma avevamo anche un altro fine, non meno importante: quello di porci come soggetto istituzionale e politico forte, ragionante e determinato, una forza tranquilla. Lo abbiamo ritenuto indispensabile dovere di fronte alle ansie e alle paure che nel Paese ci sono e che - occorre che qualcuno lo dica con chiarezza - non sono certo il frutto delle misure contenute in una finanziaria non ancora approvata, ma vengono da un quadro di incertezze e di difficoltà riconducibili in gran parte alla responsabilità del precedente Governo.

Presidente. Non mi turbano affatto. Non c'è nessuno in quest'Aula che non conosce la pericolosa deriva dell'insicurezza collettiva e credo che nessuno in quest'Aula se la possa augurare. Per questa ragione, per quell'autonoma decisione politica, per quel lavoro, il nostro voto favorevole non è un tributo esatto a scadenza dal Governo Prodi, ma è, al contrario, il frutto della frutto della qualità della relazione politico-istituzionale tra il Gruppo dell'Ulivo e il Governo, una risorsa preziosa che dobbiamo essere in grado di consolidare e di apprezzare ogni giorno. senatore Schifani, nemmeno quando interveniva il presidente Matteoli e neanche quando interveniva alcuno dei colleghi dell'opposizione, fosse o non fosse chi ritenete voi il più o il meno importante di quest'Aula, per me sono tutti

il fatto che siamo in diretta televisiva è per me grande ragione di gaudio. Siamo convinti che nessun Governo e nessun Paese sono più al sicuro se non quando le Assemblee elettive, non solo i Parlamenti nazionali, sono per davvero il luogo autonomo della rappresentanza politica, sono in grado di essere dialetticamente il lievito del saggio governare. Anche per questo, voglio porre due questioni. La prima, che è stata sollevata anche dai colleghi dell'opposizione, è quella che riguarda le regole. Ci torneremo, ma voglio qui assumere, come prioritaria tra le altre, la questione della riforma della disciplina della manovra di bilancio nei termini e con la forza con la quale il presidente Morando l'ha posta in quest'Aula. Ringrazio il presidente Morando, così come ringrazio il relatore per il lavoro di questi giorni. La seconda è quella dell'attuazione del programma, rispetto alla quale, ministro Padoa-Schioppa, questo Gruppo mette da subito a disposizione la propria incalzante forza, la propria autonoma capacità di proposta. Infine, colleghi dell'opposizione (questo vi interessa e quindi immagino che tacerete), non intendo in alcun modo - e non l'ho fatto neanche ieri - eludere la questione relativa all'emendamento in materia di prescrizione dei giudizi innanzi alla Corte dei conti... quella che ironicamente il presidente Berlusconi, che è cultore della materia, ha definito norma *ad personam*. È stato un errore grave, molto grave. Da presidente del mio Gruppo, me ne assumo intera la responsabilità, ma insieme il merito di avere chiesto immediatamente lo stralcio di quella norma... la cui presenza nel testo, lo voglio ricordare, è stata denunciata in quest'Aula per primi da due senatori del mio Gruppo, il senatore Salvi e il senatore Manzione,

davanti agli italiani. Vorrei ancora dire ai colleghi di Forza Italia che per comprensibili esigenze di polemica politica hanno ritenuto di impedire la dichiarazione di inammissibilità di quella norma (che peraltro, lo sappiamo, è in violazione della legge di contabilità dello Stato), che a questo punto è molto sottile il limite che separa l'esigenza più che legittima della polemica politica

Infine, siamo convinti che questa finanziaria sia necessaria e utile per il Paese e siamo convinti che dalla politica della palude del grave dissesto dei conti pubblici, stia nascendo il terreno compatto dal quale partire del senatore Asciutti)*. Per questo, i senatori e le senatrici del mio Gruppo passeranno davanti al banco della Presidenza e diranno «sì», per convinzione, per onorare l'impegno che l'Ulivo aveva assunto con i propri elettori, per ragionevole fedeltà al nostro Governo, ma prima di questo in celebrazione del prestigio, della responsabilità del ruolo di parlamentari della Repubblica e di dirigenti politici.

Senatori, la Presidenza non ha dato la parola al senatore Barbato mentre entrava, perché non era presente in Aula.

se siamo al punto di dover confermare nuovamente la fiducia al Governo Prodi, evidentemente non vi è stata concordia, non già nella maggioranza, bensì negli intenti di sfida ancora molto presenti tra le forze politiche attuali. Sull'auspicata cautela dei lavori di analisi del provvedimento in oggetto, è prevalsa purtroppo la caparbietà di una concezione minore di arte del governo, tutta protesa al contraddittorio fine a se stesso, piuttosto che all'alto senso di responsabilità politica. Lo scendere ancora una volta nello scontro fine a se stesso ha svilito l'impegno profuso dalla maggioranza nella valutazione del testo economico, nonostante le incessanti fatiche della Commissione. Questa fiducia mi angustia non tanto perché strumento necessario di una maggioranza stringata, ma perché ancora una volta ha significato perdita del primato della democrazia e della vera politica.

alle dichiarazioni di voto, avevo comunicato che il Governo ha fatto pervenire alla Presidenza, per il coordinamento del testo, alcune indicazioni che il senatore D'Andrea ha verificato anche con gli esponenti dell'opposizione.

della Presidenza del Senato, ha evidenziato la necessità di apportare alcune correzioni, in ordine alle quali, come lei ha già ricordato, sono stati contattati i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione. Procedo rapidamente. Al comma 1, con riferimento al saldo netto da rifinanziare, le cifre: "9.520 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.520 milioni di euro".

con le seguenti: "8,5" e "5". Al comma 1018, dopo le parole: "un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro" euro" sono inserite le seguenti: "a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009" Al comma 1193, secondo periodo,

"1325-*bis*. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009" al fine di dare senso alla norma contenuta in tabella A. Vi sono poi delle correzioni di carattere meramente formale o di coordinamento che sono già state distribuite ai responsabili dei Gruppi e che chiedo alla Presidenza, a nome del Governo, di depositare agli atti del Senato ai fini del recepimento nel testo dell'emendamento 1.1000, così come delle correzioni precedentemente analiticamente indicate. Queste sono le indicazioni concordate con gli esperti di tutti i Gruppi.

Non è possibile: questa è la cosa più scorretta che si possa fare in un'Aula, non ce n'è una peggiore! Esprimere commenti al voto di un collega, ripeto, con applausi o commenti diversi. Vi prego, senatori!

Non è accettabile, vi prego di riflettere! Non lo dico più, ma veramente vi prego di riflettere.

Bobba, Boccia Antonio,

Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai Nania ,

Colleghi, per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo dovrà ora procedere alla presentazione della conseguente Nota di variazioni, che sarà deferita alla 5a Commissione permanente. *(Vivaci

Il senatore Ciccanti, secondo il resoconto stenografico, nella seduta odierna ha detto: «Il senatore Salvi addirittura indica un potente Ministro di questo Governo quale beneficiario della norma, perché inquisito per danni patrimoniali quando era sindaco di Roma». Vorrei restasse a verbale che non ho mai detto e nemmeno pensato che sia beneficiario di questa norma l'onorevole Rutelli o alcun altro parlamentare o esponente politico di questo Governo.

dei deputati. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Terza Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007

con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge del bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge finanziaria.

la Terza Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007-2009 recepisce gli effetti dell'emendamento 1.1000 del Governo,

durante la seconda lettura del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nel quale sono stati già considerati, mediante altra apposita Nota di variazioni, gli effetti della prima lettura. Sotto il profilo finanziario, per l'anno 2007, il saldo netto da finanziare iniziale, stabilito dopo la prima lettura in 22,995 miliardi di euro, diventa pari a 22,973 miliardi di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, per effetto del differenziale fra entrate finali, pari a 26,931 miliardi, e spese finali, pari a 39,451 miliardi. Vengono, in tal modo, recepiti gli effetti della manovra sul bilancio dello Stato in termini di competenza per 23 milioni di euro. Le variazioni contenute nella Nota in esame comportano quindi modifiche all'allegato n. 1 al disegno di legge di bilancio, relativo all'elenco delle unità previsionali di base, ai quadri generali riassuntivi per l'anno 2007, in termini di competenza e di cassa, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009, in termini di competenza, nonché al bilancio programmatico. Infine, vengono apportate modifiche allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di tutti i Ministeri. Verificata pertanto, signor Presidente, la rispondenza della Nota di variazioni al contenuto della manovra finanziaria appena approvata, invito quest'Aula al voto favorevole alla Nota di variazioni e al disegno di legge n. 1184 recante il bilancio di previsione dello

il dato politico è che avete aumentato le tasse per far pagare quasi 1 miliardo di euro di spese in più, e questo già lo abbiamo detto. In questo modo otteniamo un miglioramento del saldo netto da finanziare da 23 miliardi, mentre per quanto riguarda la cassa otteniamo un peggioramento di 77 espresso al netto delle regolazioni debitorie. Se invece guardiamo al lordo delle regolazioni debitorie, troviamo un peggioramento di circa 3 miliardi per la competenza e di 4 miliardi per la cassa. Ciò non quadra, però, con i dati relativi

un saldo netto che viene modificato per 33,7 miliardi, mentre il fabbisogno e l'indebitamento per una cifra, stranamente coincidente, di 29,6. Quindi, mentre per la Nota di variazioni si registra un risultato di competenza migliore rispetto a quello di cassa, ciò non avviene, e per valori molto alti, per quanto riguarda le spese toccate nella finanziaria. Ho posto questa domanda in Commissione, ma il rappresentante del Governo non mi ha risposto: non so se non ha voluto o non è stato in grado. In quest'Aula è presente ora il Ministro dell'economia e credo che possa - chi meglio di lui? - dare al Parlamento una risposta chiara su una questione che non è banale perché, se i dati tra la Nota di variazioni e la copertura della finanziaria variano per un'entità così grande e, soprattutto, è diverso il segno della competenza e della cassa,

il Governo ha detto che l'ultima Nota di variazioni apportata era sui dati di settembre e che non vuole incorporare nel bilancio di previsione l'andamento delle maggiori entrate emerso l'11 dicembre. dicembre. Quindi, per prudenza, il Governo non mette in questo bilancio 25 miliardi di maggiori entrate realizzate già nel 2006. Come ho già detto, a mio parere, anche se non c'è una norma

trasposizione della legge finanziaria nella legge di bilancio, in modo che diventi esecutiva per l'esercizio prossimo, non posso non ricordare, entrando

Questo vuol dire - voglio ricordarlo a tutta l'Aula - che la differenza è stata di cinque voti, guarda caso il numero dei voti dei senatori a vita.

risulta in quest'Aula che i parlamentari liberamente eletti dal popolo italiano hanno negato la fiducia al presidente Prodi e al suo Governo e che

per favore. Capisco che la coscienza sporca di qualcuno impedisce di accettare queste semplicissime parole che io ribadisco, sperando che la coscienza di qualcuno possa valutare attentamente quanto ho detto e che ripeto: oggi

tra l'altro, non ritengo vi sia altro da aggiungere sul significato politico della votazione precedente: una fiducia concessa con una maggioranza di alcuni parlamentari, privi di suffragio elettorale e quindi anche politico. Sta al Paese interpretare il significato di questo voto, la forza di questo Governo, come esce da questa finanziaria e da questo voto! Avevo chiesto di intervenire e la ringrazio per avermi dato la parola. Ho ascoltato con attenzione l'intervento dei colleghi che si occupano più dettagliatamente del sottoscritto della tematica della finanziaria, della Nota di variazioni e del voto sul bilancio.

per un artifizio contabile che vogliamo disconoscere e delle cui ragioni preferiamo essere tenuti all'oscuro, dato che si sta realizzando un falso contabile in contabilità pubblica. Alla luce di tali considerazioni, riteniamo di manifestare il nostro dissenso in un modo diverso, non diverso, non partecipando al voto, perché riteniamo di non poter contribuire alla votazione su un falso contabile.

di esprimere un voto, sostenendo che in questo bilancio ci sono implicazioni di falsità e nonostante questo, per carità, il Senato lo ha approvato; quindi, legittimamente rispettiamo il voto sulla legge finanziaria.

allora smentito il suo intervento, perché egli ha affermato che in questa finanziaria non ci sono nuove e maggiori spese correnti, anzi che c'è un risparmio delle spese correnti. Quindi, il bilancio è falso e noi,

Il voto che è stato espresso poc'anzi è legittimo. Non dirò mai che non è un voto legittimo, però il risultato porta ad un voto di

però questo è ciò che fa la differenza. E allora, se un senatore dell'opposizione prende la parola per mettere in rilievo questo aspetto politico, credo sia legittimato a farlo, ha il diritto di farlo; chi non lo vuole ascoltare può essere dall'Aula ma non si può consentire che qualcuno tenti addirittura di aggredirlo perché sta facendo una denuncia politica in quest'Aula. Questo non è assolutamente consentito Matteoli, per la verità, la reazione vivace c'è stata, un tentativo di aggressione non mi pare. Comunque, qui dentro tutti hanno il diritto di parola e di fare discorsi politici anche forti.

non ha visto che, poc'anzi, ho avuto modo di avvicinarmi al banco del senatore Cossiga, con il quale, senza insulti, ho manifestato una mia opinione.

vorrei un attimo di attenzione dai colleghi, anche dell'opposizione. Signor Presidente, noi abbiamo iniziato una legislatura molto difficile, una legislatura molto difficile, perché segue una legge elettorale che ha condizionato la composizione del Parlamento. legge elettorale aveva nelle intenzioni esplicite e dichiarate che tutti abbiamo potuto leggere sui *media*...

di evitare che vi fosse un'unica maggioranza nei due rami del Parlamento. *(Commenti del senatore Storace).* La legge elettorale voleva determinare le condizioni per cui la Camera avesse una maggioranza e il Senato ne avesse un'altra.

fermi qui, ascoltando insulti da parte di un'opposizione che non consente al Parlamento di lavorare. Questo, signor Presidente, è inaccettabile. Noi non possiamo... PRESIDENTE. Adesso è stato lei a uscire fuori dal seminato. Oggi questo Parlamento ha lavorato e funzionato in maniera egregia fino a dieci minuti fa;

con qualunque sistema elettorale, quando il corpo elettorale esprime due giudizi diversi, si avrebbero una Camera ed un Senato con maggioranze diverse. Il sistema elettorale vigente in Italia ha avuto soltanto, ahimé, una funzione: di fare in modo che, nonostante la nostra maggioranza nel Paese, voi aveste una maggioranza in Parlamento, anche se molto più limitata che alla Camera.

Sto per dire una cosa a vostro favore! Signor Presidente, non vorrei fare il saputo, anche perché sono stato Presidente di questa Assemblea prima di lei,

pareva che, nel momento in cui lei ha dato la parola al presidente emerito Cossiga, ci fosse il Ministro dell'economia in piedi già col microfono acceso. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Devo dire che capita raramente di vederlo in quest'Aula: per me è la prima volta. Non credo che possa esser stato sufficiente il richiamo del presidente Cossiga

Quando ho ascoltato la sua replica, ho avuto l'impressione che parlasse di un'altra finanziaria e ho ascoltato tutto il suo intervento. Questo mi fa pensare che lui non sappia rispondere e, quindi, si deve dimettere!

Quello che è successo poc'anzi è un fatto increscioso per il Senato, per il nostro ruolo e per la nostra dignità. Il Ministro dell'economia aveva accolto correttamente l'invito dell'opposizione a dare delle spiegazioni su fatti che noi riteniamo gravi e rilevanti. Inutile ripeterlo: vi sono dei documenti, che stanno per essere votati, che non tengono conto di un dato contabile e storico, ossia di entrate nelle casse dello Stato che non vengono contabilizzate ai fini della manovra che è stata proposta al Parlamento. Preferisco dimenticare quello che è successo, signor Presidente, perché non credo che questa scena, questa scenetta - mi si consenta la battuta - possa rimanere nella storia del nostro Parlamento come una scena da ricordare. Il Ministro si è alzato, poi gli è stato quasi ingiunto da un altro collega o da altre persone della sua stessa maggioranza, con gesti eclatanti, di non parlare. Signor Presidente, noi in questo Senato lavoriamo poco:

siamo portati ad approvare pochissime leggi, a votare pochissimi emendamenti proprio per la paura del Governo di andare sotto. Siamo abituati alle fiducie - è la decima in sei mesi - e quindi questo ramo del Parlamento è stato svuotato della sua funzione.

che non fanno onore al ruolo del parlamentare. Non avvicinatevi più al banco del Governo a fare segnali: così non si parla, non parlare. Il Ministro è autonomo, ha la sua dignità, la sua autorevolezza; la spieghi, la dimostri, risponda alle nostre richieste! Non verrà lapidato, verrà rispettato perché noi rispettiamo, le istituzioni.

che ha avuto la sensibilità di chiedere la parola per rispondere a delle sollecitazioni di molti colleghi dell'opposizione e ha subito una vera e propria intimidazione da parte di alcuni colleghi della sua stessa maggioranza. Credo che un episodio del genere non abbia precedenti nella storia del Parlamento italiano. (*Richiami del Presidente).* Non ho finito, signor Presidente. Vorrei che lei spiegasse all'Assemblea per quale motivo, nel momento in cui il Ministro dell'economia ha chiesto la parola e stava per parlare, il presidente Cossiga ha avuto la parola per intervenire al posto del Ministro dell'economia. Vorrei capire per quale motivo ha impedito al Ministro dell'economia di prendere la parola per rispondere alle nostre sollecitazioni. *(Applausi dal Gruppo AN).* PRESIDENTE. Signor Ministro, la parola a lei,

La parola non mi è stata data, o mi è stata tolta, perché è stata sollevata una questione di procedura, e cioè - se ho capito bene - è stato detto...

Penso che la decisione se riaprire o no il dibattito, signor Presidente, spetti a lei e non a me. COSSIGA

Sarà poi lei, Presidente, a decidere se il dibattito si riapre o no. Io rispondo sulla questione che è stata posta. Premetto che, se il mio intervento è stato ascoltato, esso contiene le risposte a quasi tutte le domande che sono state fatte, in particolare a quelle del senatore Baldassarri. BALDASSARRI *(AN)*. Dove? MORANDO *(Ulivo)*. L'attuale Terza Nota di variazioni recepisce gli effetti finanziari differenziali, derivanti dall'approvazione della proposta di legge finanziaria, così come approvata al Senato rispetto alla Camera. Per quanto attiene all'andamento delle entrate tributarie, il Governo ricorda che l'assestamento al bilancio, presentato al Parlamento lo scorso settembre, ha recepito le maggiori entrate.

Infine, per quanto attiene alla differenza della Nota di variazioni per l'anno 2007 espressa in termini di competenza e di cassa, si tratta dei 100 milioni di sola cassa iscritti nel fondo per la compensazione degli effetti derivanti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali, che passa da 420 milioni a 520 milioni. Grazie.

Signor Presidente, nella mia dichiarazione

essendomi limitato ad indicare e riferire un colloquio tra giornalisti e alcuni colleghi senatori, tra cui il senatore Salvi, riportato da una nota dell'agenzia AGI di ieri, 14 dicembre.

ma solo una valutazione politica che, se è sbagliata, basta che sia chiarita ed argomentata. Dal momento che per principio credo alla buona fede di tutti, non ho alcun dubbio sulla buona fede del senatore Ciccanti. Mi limito a ricordare che nell'intervento di questa mattina egli ha detto testualmente: «II senatore Salvi addirittura indica un potente Ministro di questo Governo quale beneficiario beneficiario della norma perché inquisito per danni patrimoniali quando era Sindaco di Roma». Dal momento che non c'è alcun altro Ministro, potente o non potente, in questo Governo che sia stato Sindaco di Roma, era del tutto chiaro - così è stato inteso - il riferimento all'onorevole Rutelli. Del resto, la la nota di agenzia citata è di assoluta chiarezza. Al giornalista che chiedeva: «Non c'è qualche altro ex Sindaco di Roma che aveva qualche problema?», Cesare Salvi non aggiunge altro e risponde: «Non faccio dietrologia».

un dibattito sulla situazione del Medio Oriente e, in particolare, del Libano nel quale sono impegnati migliaia di nostri soldati. Da parte sua, Presidente, c'era stata un'iniziativa nei confronti del Governo che, secondo quanto da lei comunicato,

diverse settimane. Speriamo dunque che in questo frangente non accada qualcosa rispetto a cui sarebbe stato bene essere preparati da una doverosa relazione del Governo al riguardo.